finestra"). Comunico che, in data 20 giugno 2017, è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno:* «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»

si riunisce esattamente ad un anno di distanza dal *referendum* britannico che si tenne il 23 giugno dello scorso Doveva essere un anno orribile per l'Europa, per l'Unione europea e le previsioni non sono state del tutto rispettate. Viviamo in un clima certamente complicato, ma molte delle previsioni di quelle settimane si sono rivelate infondate. Un anno fa l'Unione europea era, in effetti, al centro di una sorta di tempesta perfetta a causa dell'uscita di un Paese fondamentale come il Regno Unito, si potrebbe dire un Paese dall'europeismo riluttante, un Paese che non aveva naturalmente aderito all'euro, ma tuttavia un protagonista della storia e dell'economia

l'edificio europeo - che nel corso dei decenni era andato via via crescendo dai sei Paesi fondatori sino ad arrivare ai 28 - per la prima volta vedeva un membro, di questo peso e di questa influenza, decidere di uscire. l'impatto di questo *referendum*, la crisi migratoria, gli effetti della crisi economica più grave del dopoguerra e il conseguente diffondersi, se andiamo a rivedere lo stato d'animo della discussione pubblica in Europa, non solo di non solo di uno scetticismo verso il progetto europeo che, con maggiore o minore forza c'è sempre stato nel corso dei decenni, ma di una vera diffidenza o addirittura ostilità,

la risposta ai nostri problemi ma, in un certo senso, ne era l'origine, la causa di tutti i mali, il bersaglio di tutte le critiche. Ebbene, un anno dopo ci troviamo di fronte a uno scenario diverso. Lunedì sono cominciati formalmente i negoziati successivi all'attivazione dell'articolo 50 dei Trattati per l'uscita del Regno Unito e sono iniziati in un clima in cui certamente chi ha deciso di uscire non si presenta al tavolo negoziale con una forza contrattuale particolare. Voglio dire qui, per inciso, tra l'altro, che la posizione italiana non è favorevole - visto che c'è una discussione di questo genere in Europa - né ad una *hard* Brexit né ad una *soft* Brexit. Penso che abbiamo bisogno di condurre questo negoziato con l'obiettivo di una chiarezza nei rapporti tra un Paese così importante e l'Unione europea, e che, per parte italiana, dentro questa chiarezza, deve esserci in particolare chiarezza sui diritti e sul destino delle centinaia di migliaia di nostri concittadini che risiedono nel Regno Unito. Certo, il modo in cui comincia quel negoziato è un segno di come le cose sono andate evolvendosi in questo anno. Insomma, si potrebbe dire che Brexit, quella decisione imprevista, e per certi versi storica, più che una campana a morto per il progetto

il voto inglese, più che come l'inizio della fine del progetto dell'Unione, come un campanello d'allarme che ha rimesso il progetto dell'Unione al centro della discussione pubblica nel nostro continente. Diciamo almeno una cosa: il progetto dell'Unione, proprio nel suo momento più critico, di quella tempesta perfetta cui accennavo prima, ha confermato la propria vitalità: resta un progetto centrale per il nostro futuro. Nei giorni scorsi abbiamo ricordato la figura di un grande cancelliere tedesco, cristiano-democratico, Helmut Kohl, alla cui memoria credo debba andare anche l'omaggio del Senato della Repubblica. *(Applausi dai

della pacificazione, dello sviluppo economico; è stato il secolo del superamento delle dittature nel blocco dell'Est, della riunificazione tedesca, dell'avanzata del percorso europeo. In questo, Helmut Kohl ha avuto un ruolo fondamentale. Sarà difficile dimenticare quell'immagine della lunghissima stretta di mano tra Kohl e Mitterand al cimitero di Verdun.

dicendo che gli spiriti del male non sono stati banditi per sempre dall'Europa; a ogni generazione si pone di nuovo il compito di impedire il loro ritorno. Bene, ora questo compito è il nostro, è il compito di chi governa, di chi ha responsabilità politiche e di chi ha responsabilità in generale nelle nostre società. Ora che si riscopre la vitalità del progetto, resta attuale il compito di bandire gli spiriti del male, che hanno portato a quella prima parte del Novecento che non possiamo dimenticare. E con orgoglio io rivendico il fatto che questa vitalità del progetto europeo è stata incoraggiata e in parte anche, se volete, scoperta proprio qui a Roma, nel mese di marzo, nell'occasione di quella dichiarazione comune per i sessant'anni dei Trattati di Roma, dei Trattati dell'Unione. Non è stato un successo del Governo: è stato un successo del Paese, della città, del significato simbolico che questa città e questo Paese hanno avuto nella storia e nella costruzione del percorso europeo. Ora abbiamo questa responsabilità, ora che l'Unione, superpotenza tranquilla (come qualcuno l'ha definita), ha uno spazio geopolitico maggiore di prima, semplicemente per il fatto che il nostro principale alleato, che naturalmente resta il nostro principale alleato, cioè gli Stati Uniti, ha adottato una linea che lo vede più concentrato sulle dinamiche e sulla dimensione interna e sugli interessi economici del proprio Paese, apparentemente, almeno in questa fase, meno proiettato sul piano politico politico e commerciale sugli scenari globali. La superpotenza tranquilla ha uno spazio da riempire, dal punto di vista geopolitico, che la interpella. Ora Ora abbiamo in parte sulle nostre spalle (non da soli, perché non c'è solo l'Unione europea), il compito di tenere aperta la strada conclusa con gli accordi di Parigi nel dicembre 2015, che porta a contrastare il cambiamento climatico, secondo una linea che abbiamo condiviso immediatamente con il presidente Macron e con la cancelliera Merkel, poche ore dopo la decisione formale, annunciata dagli Stati Uniti, di non riconoscersi più negli accordi di Parigi, secondo la linea che con Merkel e Macron abbiamo affermato della non negoziabilità di questi accordi. accordi. Dire che non si rimettono in discussione significa dire che non si rimettono in discussione. So benissimo che l'intenzione degli Stati Uniti non è quella di negare il tema del cambiamento climatico, ma è quella di ridiscutere gli impegni economici che i grandi Paesi, i Paesi più ricchi e le aree del mondo più sviluppate, hanno messo sui fondi per il contenimento degli effetti del cambiamento climatico a favore dei Paesi più poveri. Ma proprio di questo si è trattato quando si è trattato di negoziare COP 21 a Parigi ed è proprio questo che noi non intendiamo rinegoziare. Ora quindi abbiamo la responsabilità di portare avanti Naturalmente, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, il Governo non ha alcuna intenzione di passare da una fase, che forse c'è stata in qualche parte della nostra opinione pubblica, di demonizzazione dell'Unione europea a una fase di euforia o acritica esaltazione del progetto europeo. europeo. Il progetto dell'Unione certamente è più che mai attuale, ma l'Unione deve cambiare. Noi dobbiamo avere l'orgoglio e il coraggio di tenere assieme questi due elementi, cioè di dire con forza che ci riconosciamo nel carattere strategico del progetto dell'Unione, ma che al tempo stesso, perché questo carattere strategico sopravviva, cresca e si sviluppi, c'è bisogno di cambiare. L'edificio dell'Unione ha bisogno di essere cambiato. Mi auguro che questa missione possa essere rafforzata anche dalla nuova *leadership* francese che ha giocato una parte della campagna elettorale che ha portato il presidente Macron a un successo così significativo proprio sul tema della scommessa sull'Unione europea e sul suo cambiamento. La crescita dell'eurozona è migliore del previsto, a maggior ragione, che la crescita non può essere soffocata da regole che sono state concepite in un periodo diverso, in un'epoca di crisi e difficoltà in cui sarebbe stato molto audace e difficile immaginare una crescita europea del 2 per cento, quella che va profilandosi nel 2017 e negli anni seguenti. crescita ha bisogno di una vera unione monetaria, di politiche del lavoro e degli investimenti. Insomma, non bastano i numeri e non bastano i decimali. Europa significa lavoro, *welfare*, inclusione e crescita: è questo che ha determinato il successo del modello europeo, sia nei nostri Paesi che in quelli che sono entrati in Europa, e che determina oggi la sua capacità di attrazione a livello internazionale. O noi scommettiamo su queste caratteristiche dell'Europa libera, democratica e sociale oppure faremo fatica, dopo questa sveglia che è venuta negli ultimi mesi, a continuare a investire, a rafforzare e a far crescere il progetto comune. Ne parleranno a metà luglio a Roma i Ministri dell'economia di Francia, Germania e Italia. Per noi questo resta l'impegno fondamentale: lo diciamo da anni e ci auguriamo di dirlo sempre più in buona compagnia, affinché non sia più soltanto una battaglia italiana, o considerata una battaglia di alcuni Paesi economicamente più in difficoltà, ma diventi una battaglia europea

il Consiglio di domani e dopodomani si concentrerà in particolare su due questioni: la prima è la questione della sicurezza e della difesa,

spingono i Governi e l'Unione a essere più attivi e presenti sul terreno della sicurezza. Gli orribili attentati che hanno colpito Manchester e Londra che ieri, sia pur fallito, ha colpito di nuovo Bruxelles, dove si incontrerà il Consiglio europeo, ci dicono che la minaccia è comune e ha bisogno di risposte comuni. Queste risposte, che hanno a che fare da un lato con il controllo e dall'altro con la riduzione del fenomeno della radicalizzazione collegata al fondamentalismo islamico, da cui nascono le minacce terroristiche, va contrastato va contrastato a livello europeo su due piani. Da un lato, certamente perfezionando - e il Consiglio europeo se ne occuperà - alcune misure molto specifiche di scambio di informazioni sui viaggi e sugli ingressi e le uscite sul territorio europeo; dall'altro - e finalmente, dico io - anche sulla scia di quella dichiarazione di Taormina che il G7 ha emesso un mese fa, cercando di moltiplicare la pressione (e finalmente di ottenere anche qualche risultato) sui grandi *player* del *web* nei confronti dei fenomeni di radicalizzazione. possono essere individuati e contrastati da chi detiene le chiavi di un numero così impressionante di dati, in un contesto così globale come quello dei *social network*. network*. La rete, che è lo strumento della nostra libertà, non può diventare il terreno di coltura della minaccia alla nostra sicurezza. proposito, la dichiarazione di Taormina sarà ripresa dal Consiglio europeo di domani e dopodomani e credo che noi dobbiamo essere - con tutto il rispetto per la libertà d'impresa molto esigenti nei confronti dei grandi *player* di Internet. Non è possibile, infatti, che noi coltiviamo, attraverso questo magnifico strumento di libertà, la minaccia alla nostra sicurezza. *(Applausi compirà nel Consiglio di domani e dopodomani - e noi ci batteremo per questo - un ulteriore piccolo passo in avanti (si procede per piccoli passi ed è inutile

la Commissione ha proposto un fondo comune per la difesa europea. Il suo presidente, Juncker, ha parlato della possibilità, attraverso questo fondo comune per la difesa, di risparmiare tra i 25 e i 100 miliardi di euro, a seconda dell'intensità e del ritmo con cui si lavorerà in questa direzione nei bilanci dei diversi Paesi sulla difesa. quindi, parlando di una cosa importante, non solo, come è ovvio, dal punto di vista geopolitico (la superpotenza tranquilla, che occupa uno spazio geopolitico che può essere lasciato vuoto e che ha bisogno di essere occupato, perché gli spazi

il Governo, assieme ai Governi degli altri tre grandi Paesi europei, in un incontro a Versailles tra i quattro Capi di Governo di Italia, Spagna, Francia e Germania,

Ebbene, quell'idea fu lanciata esattamente nell'incontro di quei quattro Capi di Stato e di Governo a Versailles e aveva al centro l'obiettivo della difesa comune; la difesa comune come terreno sul quale questa Europa a diversi livelli di integrazione, senza modificare i trattati, può fare dei passi in avanti e credo debba farli.

che, nonostante qualche passo in avanti, la velocità con la quale l'Unione europea si muove sul terreno delle politiche comuni per l'immigrazione resta drammaticamente al di sotto delle esigenze di governo e di gestione di questo fenomeno. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo e lo diremo apertamente anche a Bruxelles. Certo, Certo, si potrebbe rivendicare che si è ottenuto qualche risultato, almeno sul terreno simbolico. Proprio in quest'Aula avevo parlato alcuni mesi fa del fatto che per l'Italia era inaccettabile l'idea di una sorta di Europa a due diverse rigidità. Una rigidità totale, assoluta, massima, quando si trattava di affrontare questioni relative a regole di bilancio e una rigidità totalmente flessibile, flessibile, quasi inesistente, quando si trattava di rispettare gli impegni comuni sul terreno dell'immigrazione. Non potevamo accettare questa idea e a me fa piacere che la Commissione europea abbia annunciato, una settimana fa, l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti di quei tre Paesi europei, che, in modo esplicito, avevano dichiarato di non voler accettare gli impegni, che pure erano stati sottoscritti dal Consiglio europeo, che dovrebbe essere impegnativo per tutti. Credo però che non ci possiamo consolare con questa soddisfazione morale, che certamente darà un contributo, almeno in parte. Abbiamo bisogno di andare molto più rapidamente verso una politica comune; penso alla politica comune che l'Italia ha proposto nei confronti dell'Africa.

si deve fare di più nei confronti degli sforzi che l'Italia ha messo in campo in rapporto con la Libia. Abbiamo aperto una strada: lo voglio dire molto apertamente alle senatrici e ai senatori. Lo abbiamo fatto anche prendendoci le nostre responsabilità come Paese, nell'aprire un'ambasciata, nello stipulare degli accordi con un Governo la cui fragilità si conosce perfettamente, nello stipulare accordi con le tribù che controllano la parte meridionale, al confine con il Niger, nell'investire su questi accordi e nel lavorare per rafforzare la guardia costiera, che fa capo al Consiglio presidenziale guidato dal presidente Serraj,

Dalla guardia costiera libica, infatti, che fa capo al Consiglio presidenziale, sono state recuperate alcune migliaia di migranti nelle ultime settimane: è un fatto nuovo, che non dobbiamo "sbandierare" o esaltare troppo, ma che ci indica che una strada è stata aperta. Quello che vogliamo sapere dall'Unione europea è se, su questa strada che l'Italia ha aperto, c'è l'Unione europea alle nostre spalle, con le sue risorse e con il suo impegno politico, o se dobbiamo continuare a cavarcela da soli. L'Italia è in grado di gestire tale questione, sia pure con difficoltà crescenti, che al Governo non sono certamente sconosciute, ma l'Europa, se vuole recuperare la sua vitalità, se vuole cambiare, se vuole scommettere sul proprio futuro, oltre ad avere politiche che accompagnano la crescita, gli investimenti e il lavoro, deve avere una politica migratoria comune. Questo pretendiamo a Bruxelles e lo faremo anche nel Consiglio europeo dei prossimi giorni Infine, c'è una nota a margine nel Consiglio europeo di domani e dopodomani, che tuttavia riveste un'importanza notevole per il nostro Paese, anche se credo sarà affrontata in modo marginale, perché non si tratta di prendere decisioni, ma di discutere sui criteri; è però utile che il Senato ne sia informato. La nota a margine riguarda la decisione sui criteri da adottare per il trasferimento da Londra a Paesi dell'Unione europea principalmente di due grandi Agenzie, che attualmente hanno sede a Londra.

di avere con la città di Milano, per tante ragioni che il Senato conosce benissimo, tutte le carte in regola, non solo dal punto di vista dell'importanza della filiera farmaceutica a Milano e in Italia, ma anche dal punto di vista della qualità della vita, dell'accoglienza, della logistica, dei trasporti, della sede che potenzialmente potrebbe ospitare questa Agenzia; pensiamo di avere un *dossier* competitivo. La spinta che cercheremo di dare al Consiglio europeo - lo dico in modo semplice e penso che tra noi ci capiamo - è che questa decisione avvenga sulla base

gruppo di Paesi europei, che non farebbe certamente bene al settore di cui questa Agenzia è responsabile. Quindi noi, avendo una candidatura competitiva e forte, cercheremo di orientare la scelta in un'altra direzione.

e un gruppo di lavoro guidato dal professor Moavero Milanesi se ne sta occupando da molte settimane. È chiaro, in conclusione, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, che ci troviamo in un frangente per l'Europa di grandissimo interesse. Non c'è stato il crollo che molti avevano temuto o auspicato (a seconda dei gusti), ma non deve esserci l'illusione che l'Europa se la sia cavata, che vada bene così, che vada avanti nei binari prestabiliti. Proprio perché non c'è stato quel crollo, questo è il momento di investire per cambiare, per far crescere il progetto europeo. Un grande intellettuale inglese ha ricevuto quest'anno il premio Carlo Magno, Timothy Garton Ash, e nel riceverlo ha definito l'Europa come perennemente incompiuta e quindi - aggiungeva, forse ottimisticamente - anche sempre e per sempre giovane. Non so se sia vero che il fatto di essere incompiuta dia un dinamismo giovanile al progetto dell'Unione europea, ma so che su questo dobbiamo puntare;

se avrà il sostegno del Parlamento, naturalmente con le distinzioni ovvie tra maggioranza e opposizione, il Governo italiano in questa grande opportunità potrà svolgere il ruolo che compete a uno dei grandi Paesi fondatori.

Signora Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, desidero prima di tutto esprimere il mio più vivo apprezzamento a lei, signor Presidente del Consiglio, per la dignità con cui sta rappresentando l'Italia nel contesto internazionale, per il rispetto di cui gode, di cui a tutti noi giungono gli echi, e per l'efficacia con cui svolge questa azione. *(Applausi Con riferimento alla sua relazione di questa mattina, signor Presidente del Consiglio, devo dire che condivido sia l'analisi che le tonalità e l'impulso politico che lei le ha conferito. Vorrei toccare rapidamente tre punti, tutti di carattere strettamente politico. Quanto al primo, effettivamente, come lei ci ha illustrato, a un anno dal voto nel *referendum* britannico abbiamo visto - speriamo che continui e questo richiederà lo sforzo di tutti - una vera e propria riscossa da parte dell'Unione europea. Quello che però mi preme sottolineare è che ciò è avvenuto non solo ad opera dei responsabili dei Governi degli Stati membri, molto più uniti di quanto si potesse immaginare anche nel modo di affrontare il negoziato con il Regno Unito.

per l'uscita di quel Paese: conseguenze in quel Paese, dalla *disruption* del sistema politico‑amministrativo, alla totale incertezza in cui il Regno Unito, purtroppo per tutti noi (oltre che per loro), è piombato. Questo si riflette in quella che potremmo chiamare la prevalenza, registrata quest'anno, dell'"effetto anticorpi" rispetto all'"effetto contagio". Si temeva infatti il contagio da Brexit, Brexit ha scatenato una quantità di anticorpi, non solo nei comportamenti dei responsabili politici degli Stati, ma anche nei cittadini. in tutti i sondaggi di opinione per quanto riguarda l'aumentato - non diminuito - grado di sostegno espresso dai sondati

Questa forza viene dai Governi e dai Parlamenti. A tal proposito, vorrei suggerirle di stimolare di più il Parlamento italiano per dare questa forza. viene periodicamente a riferirci, in un modo che troviamo molto interessante (e speriamo che lei trovi interessante per il Governo gli stimoli che da qui le possono venire),

e i cinque documenti che si inscrivono nella prospettiva del Libro bianco (l'ultimo dei quali uscirà il prossimo 28 giugno e sarà sul bilancio dell'Unione europea) e che voi, Capi di Governo, nel Consiglio europeo del prossimo dicembre, dovrete trarre le conclusioni in termini di decisioni sul futuro dell'Europa. Penso, come ho già accennato in un'occasione precedente, che il Senato e la Camera debbano poter dare un contributo maggiore e più sistematico alla preparazione della posizione italiana in questo

del cancelliere Kohl e del presidente Miterrand. Su questa linea, vorrei richiamare alla memoria di tutti un gesto forse ancora più significativo da parte tedesca, stimolato da parte italiana. Era il 24 marzo del 2013, il presidente Napolitano aveva invitato il presidente federale Gauck nel luogo più difficile per un tedesco, Sant'Anna di Stazzema, dove il 12 agosto del 1944 560 civili erano stati trucidati in uno dei più orrendi eccidi. Ci fu un abbraccio tra il presidente Napolitano ed il presidente Gauck, in quello che probabilmente è stato l'ultimo atto pubblico della prima presidenza Napolitano.

portato alla memoria di tutti noi come sia stato un grande costruttore non solo di una Germania unita, ma anche di un'Europa più unita. C'è secondo me una riflessione da trarre: lo è stato perché, giunto all'apice del potere, non ha esitato a correre il rischio di perdere un'elezione, come infatti è accaduto nel 1998, a fronte di un candidato,

e l'integrazione europea sarebbe notevolmente più indietro. Signora Presidente, il Presidente del Consiglio ci ha disegnato lo scenario di un nuovo assetto globale che si è venuto delineando nell'ultimo anno e io credo che il Consiglio europeo di domani sia molto significativo, perché è il primo che si svolge dopo alcuni eventi che, nel bene e nel male, potranno insieme rappresentare il catalizzatore capace di spingere l'Europa verso una nuova fase della sua storia. Il G7 di Taormina, tenutosi dopo la vittoria di Trump e della Brexit, e la vittoria di Emmanuel Macron in Francia hanno ridisegnato le relazioni transatlantiche e hanno reso eclatante ciò che da tempo era chiaro, e cioè che l'Europa dovrà assumere sempre di più su sé stessa la responsabilità della propria sicurezza e della propria difesa e che per farlo dovrà accelerare il processo di integrazione politica ed economica. La signora Merkel, che presumibilmente continuerà a guidare la Germania anche nei prossimi anni, ne è pienamente consapevole ed il nuovo corso francese che nasce sotto il segno europeista e la figura carismatica del giovane Macron può determinare un'evoluzione delle opinioni pubbliche degli Stati europei più riluttanti. Proprio partendo da queste considerazioni, ieri Anthony Giddens, intervistato da «la Repubblica», esprimeva la certezza che l'Europa finirà per ritrovare il suo ruolo globale. Personalmente non sono però convinta, come invece sosteneva Anthony Giddens, che sarà da solo l'asse franco-tedesco a ridare la spinta in questa direzione, perché dopo la Brexit la Germania in un rapporto uno a uno con la Francia è ancora troppo più forte e e perché la Francia non riuscirebbe da sola a riorientare l'Europa verso i nuovi obiettivi che Macron ha indicato per un'Europa che voglia ritrovare la legittimazione popolare e democratica. agli obiettivi della crescita, dell'occupazione e della lotta alle diseguaglianze, da perseguire con politiche e con riforme che si facciano carico di coloro che sono colpiti o rischiano di rimanere esclusi dai processi di globalizzazione e dall'impatto della rivoluzione digitale. Innovazione e protezione. Questo è il binomio che io credo debba essere oggi la bussola delle politiche europee e di quelle nazionali. Per fare questo c'è bisogno d'Italia, di un forte asse franco-italiano; un asse che è augurabile si manifesti già dal Consiglio europeo di domani che ha all'ordine del giorno, come lei ha sottolineato e come ci ha illustrato ampiamente, alcuni dei dossier più importanti, sui quali potrà manifestarsi concretamente una rinnovata spinta europeista, pur con i tempi e la gradualità propria delle istituzioni europee. Il primo punto, forse il più rilevante, riguarda la difesa e la sicurezza europee, in ordine alle quali la bozza delle conclusioni esplicita in modo netto l'impegno ad attivare le norme del Trattato sull'Unione europea relativo alla cooperazione strutturata permanente, dando così, come lei ricordava nella sua introduzione, un seguito concreto agli impegni sottoscritti a Roma in occasione del sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma e per i quali il suo Governo e lei personalmente, signor Presidente del Consiglio, avete così intensamente lavorato. l'accelerazione verso l'integrazione della difesa europea è imposta non solo dal mutamento dello scenario globale, ma anche dalla constatazione che la Germania, per parte sua pragmaticamente e in modo molto poco vistoso, sta integrando le sue forze armate con quelle di alcuni Paesi dell'Europa dell'Est. È quindi opportuno e direi anzi indispensabile, se si vuole evitare un riarmo unilaterale (specie dopo la Brexit), che il processo cui accennavo poc'anzi si sviluppi dentro il quadro dell'Unione europea. Peraltro questo impegno, accanto a quello per l'accelerazione del programma per lo sviluppo dell'industria europea di difesa, sostenuto dall'attivazione del fondo per la difesa europea cui lei faceva riferimento, potrà avere anche importanti ricadute per l'industria italiana, specie nel settore dell'aerospazio. Al di là delle vicende che la hanno coinvolta, considero personalmente un vero peccato che la ministra della difesa francese Sylvie Goulard abbia dovuto rassegnare ieri le dimissioni, perché da

intenzioni che in ogni caso ci auguriamo verranno confermate nel Consiglio di domani. Il secondo punto al quale anche lei ha fatto riferimento come questione centrale del Consiglio dei prossimi due giorni è quello delle politiche migratorie, che per l'Italia evidentemente riveste un interesse cruciale. Su questo punto, anche se non si arriverà a determinazioni conclusive e concrete visto che i ritmi sono così lenti, cerchiamo comunque di vedere il bicchiere mezzo pieno. È infatti significativo che nella bozza di documento finale si ribadisca, come l'Italia ha sostenuto, il carattere unitario del tema e si riaffermi l'impegno a favore di un approccio globale dell'Unione europea alla migrazione. In altre parole non sarebbe accettabile, in particolare per l'Italia come per la Grecia, separare la soluzione dei singoli punti, come pure tenderebbe a fare il Gruppo di Visegrad, rinviando il tema più controverso ma per noi essenziale, cioè quello della revisione dell'accordo di Dublino, e stralciando

il documento finale ribadirà l'invito alla Commissione ad alleviare l'onere che grava sugli Stati membri in prima linea nella gestione dei rifugiati e sottolineerà che l'intera riforma del sistema europeo di asilo europeo di asilo deve trovare il giusto grado di equilibrio tra responsabilità e solidarietà e garantire la resilienza a crisi future. Questo è il punto su cui l'Europa deve mostrare di capire qual è il suo futuro, qual è il ruolo del Mediterraneo, qual è lo scenario che si presenta nel prossimo secolo nel processo Queste affermazioni, se considerate insieme alla decisione della Commissione di aprire la procedura di infrazione nei confronti dei Paesi che hanno rifiutato di accogliere la propria quota di rifugiati, segnano un mutamento di segno nell'atteggiamento dell'Europa sui temi della gestione dei flussi migratori. E questo è sicuramente un merito del Governo Renzi e del Governo Gentiloni

ma anche indicando il sentiero delle riforme per la competitività e la crescita su cui l'Italia si è impegnata negli ultimi anni con grande determinazione. Dobbiamo sostenere la ripresa dell'economia europea e per questo il pacchetto delle azioni è molto nutrito e impegnativo. Su un punto, però, l'Italia deve insistere in tutte le sedi e in tutte le forme, anche in vista di una discussione del *fiscal compact*: l'Italia dovrà battersi perché, sia sul piano interno che da parte della Commissione europea, siano rilanciati gli investimenti pubblici e privati. A questo obiettivo dovrà essere orientata la maggiore flessibilità che ciò richiede e a questo obiettivo dovrà essere finalizzato un grande piano europeo che moltiplichi l'entità e gli strumenti del piano Juncker. Perché potremo fare tutte le riforme possibili, ma senza investimenti non ripartirà la crescita, senza crescita non ripartirà l'occupazione e senza lavoro

Signora Presidente, cercherò di essere all'altezza di un impegno europeo anzitutto restando nei tempi europei. Consentitemi, in apertura di questo mio breve intervento, di associarmi alle parole del presidente Gentiloni Silveri e del presidente Monti nel ricordo di un grande europeo e di un grande amico dell'Italia, Helmut Kohl.

il presidente Napolitano sarà tra i relatori principali, come è giusto che sia. Credo che il Parlamento italiano debba un omaggio particolare a Helmut Kohl e vorrei dire che pure l'Italia gli deve un omaggio perché Helmut Kohl, nei passaggi fondamentali in cui molti teorizzavano un'Europa ristretta e chiusa rispetto alla possibilità dell'Italia di svolgere un ruolo da protagonista, ha sempre voluto difendere il ruolo essenziale del nostro Paese in Europa. Spesso vediamo i tedeschi - diciamocelo francamente - come un po' dei carnefici, considerando il richiamo costante che essi esercitano sui conti pubblici italiani e sulla politica del rigore. Bisogna cercare a volte, però, di mettersi anche nei panni altrui e capire il rapporto tra i governanti tedeschi e la loro opinione pubblica. Comunque, per quanto riguarda la moneta unica, io ricordo le confidenze di Ciampi, molto chiare in proposito: Kohl è stato determinante affinché l'Italia non fosse esclusa dal nucleo della moneta unica. È stato veramente un grande amico dell'Italia e, soprattutto, un uomo che, come il presidente Monti ha ricordato, ha saputo sacrificare anche il proprio destino politico ad un ideale più forte, che era quello dell'Europa. Dunque, il 4 luglio questo omaggio del Parlamento italiano credo sia doveroso e necessario. Il presidente Gentiloni Silveri oggi ci ha richiamato alla vitalità del progetto europeo. Credo che in termini geopolitici noi dobbiamo considerare due cose, dobbiamo considerare due cose, cioè quello che è capitato con la Brexit e con l'elezione di Trump alla presidenza degli Stati Uniti e poi dobbiamo mettere in rapporto questi due avvenimenti, che apparentemente potevano indebolire l'Europa, la vittoria di Macron in Francia e con quello che si sta profilando nello scenario tedesco, con una conferma della signora Merkel. Bene, credo che, come sempre nella storia, fatti che apparentemente potevano indebolire l'Europa hanno in realtà messo i governanti europei di fronte alle loro responsabilità: gli alibi sono caduti. Non ci si può continuare a crogiolare, ad esempio sulla difesa europea, sulla presunta freddezza inglese perché oggi l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea impone un'assunzione di responsabilità e dunque noi siamo artefici del nostro destino, lo ritroviamo interamente nelle nostre mani. Va anche considerato che Trump ha determinato della convergenza tradizionale tra Stati Uniti ed Europa (fermo restando, lo voglio dire tra parentesi, che il legame atlantico è un elemento genetico per l'Europa che nessuno nessuno può mettere in discussione e infatti nessuno vuole metterlo in discussione). Questi due fatti hanno messo i governanti europei e le opinioni pubbliche europee davanti alle proprie responsabilità. Sono convinto di una cosa e lo dico con chiarezza: le grandi linee distintive della politica, anche della politica nazionale, oggi passano attraverso il tema dell'Europa. Noi non possiamo essere "eurotimidi". Macron ha dimostrato con chiarezza, in un Paese che è storicamente scettico rispetto all'Europa,

Noi dobbiamo avere un supplemento di orgoglio e lo dobbiamo avere indipendentemente dalle posizioni politiche tradizionali che rappresentiamo in quest'Aula. C'è un filo che lega le grandi famiglie politiche europee, un filo che lega le famiglie del socialismo europeo, del popolarismo europeo ma anche altre famiglie liberali che si sono sempre identificate nel messaggio europeo. Dunque l'Europa non deve essere solo il Cerbero - a volte la posizione è scomoda ma è doverosa

Voi conoscete le mie posizioni ma non vi è dubbio che oggi stiamo subendo un'invasione molto forte e che l'opinione pubblica - tutta l'opinione pubblica - è sconcertata e facciamo fatica a gestire i flussi migratori (basti pensare alle

se questo è vero, il nesso tra la politica di sicurezza e di difesa e l'immigrazione ha una parola sola: si chiama Africa. Il tema è l'Africa: noi dobbiamo andare lì a fare una politica,

sull'euro-mediterraneo ma, in realtà, basta pensare alla destinazione di risorse nel Mediterraneo per capire che ha fatto poco o nulla. Colleghi, noi vogliamo aiutarli a casa loro, però, quando l'olio tunisino può essere commercializzato in Europa facciamo il finimondo perché dobbiamo chiudere le frontiere. Apro una parentesi e la chiudo: noi siamo a giorni alterni a criticare la politica di Trump perché disdice la possibilità di accordi commerciali con l'Europa,

non solo per la nostra politica. Apprezzo molto ciò che Alfano e Minniti stanno facendo anche nell'Africa subsahariana (perché è da lì che bisogna chiudere i rubinetti o per stabilizzare il Governo libico) ma il punto vero

purtroppo per loro e in un certo senso finalmente - da un problema che prima riguardava solo noi, oggi capiscono che bisogna andare lì a portare la cooperazione. Presidente Gentiloni lei ha illustrato un programma e noi lo condividiamo. Mai come in questo momento e come in questi anni sulla politica estera c'è una condivisione del Parlamento. Buon lavoro, siamo con lei.

Non è una questione di forma: il rispetto del Parlamento è la condizione perché il confronto tra le opposizioni e la maggioranza sia proficuo. Lei ha ragione, Presidente, quando dice che molta acqua è passata nell'ultimo anno. Le forze potenti che hanno voluto la Brexit oggi sono

critica fortemente le politiche sociali e le riforme del mercato del lavoro che sono state imposte alla Germania e all'Italia e che Macron vuole attuare in Francia. Vede, Presidente, il suo Governo ha un'occasione storica: la crisi della mondializzazione che è ripiombata su se stessa dando spazio al confronto ringhioso tra nazionalismi: Trump e Putin, Xi Jinping, Shinzo Abe e Modi. Questa crisi sembra avere in Europa un punto di caduta provvisoria innanzi tutto nella costruzione di un regime bonapartista in Francia (la definizione è di Sergio Romano, non mia). Un regime democratico, comunque - ci mancherebbe, si è votato in quel Paese - ma una forma di democrazia che i francesi non hanno conosciuto neppure sotto la Quinta Repubblica. La novità importante, però, è che le classi dirigenti francesi sono convinte oggi che la *grandeur* si possa declinare in Europa e con l'Europa. Questa è per noi obiettivamente un'occasione. L'altra novità che ha accennato nel suo intervento Mario Monti è la continuità e l'evoluzione della linea politica tedesca, del modo di declinare l'interesse tedesco in Europa. Lì, più che l'alternanza, il gioco sembra quello di un'evoluzione all'interno di un partito-regime, ed è probabile che Angela Merkel vinca

stipendi più alti agli operai tedeschi - le classi dirigenti in Germania non vogliono mettere in questione l'assetto dei due mercati del lavoro che secondo loro è fondamentale

costruire la sua politica economica e per contare in Europa durante il suo Governo saranno molto più ampi. Però, presidente Gentiloni Siveri, serve una proposta forte: in questo quadro mondiale non ci si può limitare a giocare di sponda. Questa proposta forte deve avere il coraggio non di battere i pugni sul tavolo, come fanno i guitti da avanspettacolo, ma di dire francamente a francesi e tedeschi che parte del nostro debito pubblico va ristrutturata, offrendo in cambio una politica innovativa, che non usi più *bonus* e regali di tipo elettorale che hanno fatto crescere *deficit* e debito, ma che avvii un vero risanamento, allargando la base imponibile in questo Paese. Come? Innanzitutto combattendo la corruzione, combattendo l'evasione, per cui parte importante della spesa pubblica finisce con l'alimentare, per via di tangenti, le forze intermediarie parassitarie, le forze peggiori della nostra borghesia nazionale. Questo dovrebbe essere il *deal*. E se questo fosse il contratto con l'Europa, la parola dell'Italia in Europa conterebbe, così come si avvia a contare la Spagna, che probabilmente archivierà il suo Governo di unità nazionale. Lei sa Sanchez, l'uomo con la camicia bianca, oggi sceglie l'alleanza con Podemos e cambia assetto al suo Paese, anche aprendo alle forze catalane, cosa che il Governo centralista e corrotto di Rajoy non farà mai. Ci vuole coraggio, Consiglio. Lei ha detto che il suo Governo è fragile. È vero, ma lei può fare molto. Veniamo rapidamente ai due temi in discussione nel Consiglio. Per quanto

di Donald Trump. Donald Trump in Medio Oriente sta preparando una guerra, con il suo appoggio indiscriminato all'Arabia Saudita, una guerra di sunniti contro sciiti, che potrebbe essere una guerra di proporzioni non controllabili. Stiamo molto attenti al tipo di rapporto che c'è in questo momento tra militari americani e militari russi in quello scenario (e non solo in quello). La presa di distanza da Trump non è una posizione ideologica, ma è la condizione per costruire quell'Europa di cui lei parla. Così come un'altra condizione è la fine delle sanzioni contro la Russia, non perché noi accettiamo un regime che è autoritario (democratico, (democratico, ma autoritario) e che viola i diritti civili, ma perché quelle sanzioni sono legate a un'idea della guerra fredda che ha illuso i Paesi dell'Est Europa (spostandoli tra l'altro tutti a destra, tanto che oggi rappresentano un pericolo per la stessa Unione) che che avrebbero avuto un ombrello che non ci possiamo permettere, perché l'Europa esisterà solo se sarà fortemente autonoma dalla Russia, ma anche dagli Stati Uniti. Lei ha parlato di immigrazione, signor Presidente del Consiglio, ma sa bene che la soluzione reale del problema dipende

non di solidarietà o di assistenza, ma un intervento economico di sviluppo, che è nell'interesse dell'Europa, in quel grande continente che è l'Africa. Questa è la soluzione strutturale. Concludo, Presidente. Lei ha detto che il suo Governo è fragile. Non può non esserlo, visto che il segretario del suo stesso partito ritiene di avere il diritto di occupare il suo posto, avendo vinto le le primarie. Lei però ha un grande compito: può favorire il dibattito sulle prospettive reali del nostro Paese e dell'Europa. Se lo farà, Paolo Gentiloni Silveri, nei banchi di Sinistra Italiana, forza di opposizione, troverà sicuramente un interlocutore leale. *(Applausi

come alcuni miei colleghi hanno già avuto modo di dire, lei ha una grande forza che sta propria nella debolezza del suo Governo. Certo, sui *voucher* e sulle mozioni Consip di ieri la sua maggioranza non ha fatto una bella figura. Anzi - diciamocelo - abbiamo fatto una figuraccia internazionale

è ancora in carica. Lei deve avere più coraggio nell'ambito delle riforme, signor Presidente del Consiglio, perché noi ci siamo se lei ci porta riforme che risolvono i problemi del Paese. Il presidente Casini

soprattutto lungo la rotta del Mediterraneo centrale e il trasferimento in territorio italiano dell'Agenzia europea per i medicinali, tenendo conto del fatto che Brexit produce un mutamento profondo degli equilibri finanziari italiani a causa del legame esistente tra la Borsa italiana e la *City* di Londra (*London Stock Exchange*), specie per quanto riguarda la piattaforma elettronica che regola le contrattazioni dei titoli di Stato; per quanto

che regolano i rapporti tra le diverse componenti della spesa pubblica: in modo particolare gli investimenti, la riduzione della pressione fiscale, la sburocratizzazione, l'intervento sulla malasanità e la malagiustizia e la sottostante crescita economica, dal cui maggior sviluppo può derivare una riduzione di quel rapporto grazie a una maggior crescita del denominatore. Per l'Italia - come ha detto lei - il problema più urgente è ovviamente quello di arginare i flussi migratori: «La gestione dei flussi di migranti e richiedenti asilo verso i Paesi dell'Unione» - come è scritto nella premessa del DEF 2017 «rappresenta una sfida senza precedenti che l'Europa si trova oggi ad affrontare sul terreno della libertà di circolazione delle persone, del rispetto dei diritti umani, della sicurezza dei cittadini europei. È una crisi sistemica alla quale bisogna fornire una risposta comune a a livello europeo, mediante una gestione comune delle frontiere». Questa catastrofe umanitaria diventa immane se si considera che il numero dei minori non accompagnati ha superato i 25.000 nel 2016, e siamo già quasi a 3.000 nei primi tre mesi del 2017, e che la presenza delle donne, spesso in stato interessante, contribuisce a drammatizzare ulteriormente la situazione per la particolare violenza fisica e psicologica cui sono sottoposte. Per l'Italia, signor Presidente del Consiglio, il problema è aggravato dalle sue particolari condizioni economiche: dall'essere ancora alle prese - unico Paese europeo - con una crisi economica che non è stata superata, ma che, agli attuali tassi di sviluppo - come ricordato dal Governatore della Banca d'Italia nella sua relazione conclusiva e confermato dalla delegazione del Fondo del Fondo monetario internazionale nella sua recente visita nel nostro Paese - i livelli di benessere del 2007 saranno raggiunti solo nella seconda metà del prossimo decennio, dopo vent'anni. Signor Presidente, Presidente, non le sto a ricordare la critica radicale nei confronti del *fiscal compact*, che dovete rinegoziare. Un Paese come il nostro, che presenta un tasso di disoccupazione superiore all'11 ha poco da offrire in tema di occupazione per un numero così elevato di migranti. Ne deriva l'inevitabile ghettizzazione di coloro che sbarcano sul territorio nazionale, il proliferare di attività illegali, dall'accattonaggio alla prostituzione, fino ai traffici che generano il maggiore allarme sociale tra strati crescenti dell'intera popolazione, di cui fanno parte gli stessi migranti regolari. Lei ha detto che l'Europa deve cambiare e dobbiamo avere la forza di farlo. Ha ragione, ma ci vuole una forza anche all'interno del suo Paese, con una maggioranza coesa, che non vediamo. problema le cui caratteristiche erano quelle ricordate. Di particolare importanza appare pertanto il proposito, in agenda nel Consiglio europeo, «di riformare il sistema europeo comune di asilo, compresi i principi di responsabilità e solidarietà».

i problemi che ci angustiano e che hanno bisogno di essere risolti. Siamo convinti che, con una maggioranza forte anche nel suo Parlamento nazionale, lei avrà più forza e coraggio per risolvere i nostri problemi. Auguri, Presidente. presidente Gentiloni Silveri, abbiamo ascoltato con molta attenzione la sua relazione, apprezzandone l'ampiezza, la profondità di analisi, il garbo che appartiene alla sua decisa personalità, ma soprattutto l'intento di tracciare una linea senza perdere di vista le difficoltà oggettive. Non possiamo, però, non cogliere il perdurare di una certa confusione e - direi - la pervicace volontà di glissare sul clima. Ancora in Europa stiamo al livello in cui i *leader* discuteranno delle cause profonde delle migrazioni e degli strumenti per affrontarle. Mi sembra, signor Presidente del Consiglio, che ci muoviamo come pachidermi in una situazione che richiede, invece, tempismo e rapidità, perché, mentre ragioniamo, i flussi migratori lungo le rotte del Mediterraneo centrale non si fermano, non desistono; un fenomeno che ci sta particolarmente a cuore e che ha visto il nostro Paese, specie le regioni meridionali, in prima linea; un fenomeno che spesso e volentieri è stato sottovalutato dagli altri Paesi europei. Quante volte, proprio qui, in quest'Aula, abbiamo sottolineato la responsabilità affinché ponessero in evidenza, in tutte le occasioni, l'assenza dell'Europa prima e poi la sua insufficiente risposta. Quante operazioni dispendiose e inadeguate sotto il profilo dell'accoglienza e della gestione dell'emergenza

Abbiamo spesso sentito in quest'Aula le lagnanze per delle proposte dell'Unione europea fortemente sbagliate e inadeguate al fine di gestire una crisi così imponente. I numeri a nostra disposizione, infatti, parlano chiaramente di un fenomeno che non può essere fermato, nemmeno elevando muri. Si tratta però di un fenomeno che può e deve essere gestito, guardando alla centralità della persona umana e tenendo, altresì, gli occhi bene aperti per contrastare senza mezzi termini le orrende sacche di malaffare, di sfruttamento e corruzione, che sono venute allo scoperto, il traffico illecito di persone, ma anche l'esasperazione del *business* degli aiuti umanitari, come pure le inspiegabili lungaggini nelle procedure di riconoscimento dello *status* di rifugiato e, ancora, ancora, i sistemi appositamente organizzati per favorire l'immigrazione clandestina. Temi come l'accordo di riammissione, la ricollocazione e il reinsediamento risultano oggi essere strumenti fortemente burocratizzati, farraginosi, inefficaci e insoddisfacenti. Allo stesso modo è assolutamente necessario riformare il sistema europeo comune di asilo. Conosciamo infatti gli aspetti controversi legati alla Dichiarazione UE-Turchia, in forza della quale per l'Unione europea è possibile operare espulsioni verso la Turchia, che comunque non è da considerare un "Paese sicuro" per i richiedenti asilo, nella vigenza della regola del cosiddetto programma "uno a uno", per la quale, per ogni siriano in posizione irregolare che l'Unione europea espelle verso la Turchia, questo Stato invierà un altro rifugiato siriano in Europa. Questo programma ha sollevato delle problematiche giuridiche serie, poiché discrimina fra siriani e richiedenti asilo di altre nazionalità ed è moralmente discutibile, nella misura in cui genera una sorta di "commercio" di esseri umani. Insomma, signor Presidente, si impone un cambio di marcia serio e ci auguriamo che il Consiglio europeo dei prossimi giorni ne senta la necessità, anche se ci consentirà di nutrire una qualche sfiducia in merito. sono però solo le guerre e le migrazioni a preoccupare, ma anche l'economia mondiale. L'Europa dell'*austerity*, della moneta unica, del rigore tetragono ha mostrato tutti i suoi limiti. Questo tipo di politica non funziona: non funziona ovviamente dal punto di vista dell'economia reale, come dimostrano i dati sulla crescita del PIL; ma non funziona neppure da un punto di vista squisitamente finanziario. A cosa serve l'imposizione di tutti questi sacrifici, se poi il debito pubblico cresce in misura ben maggiore rispetto ai risparmi che si possono ottenere? Che dire poi delle asimmetrie che caratterizzano i diversi Paesi dell'eurozona? Signor Presidente, vi sono divergenze insopportabili e non è ammissibile che in alcuni Paesi la disoccupazione sia ai minimi storici, mentre in altri Paesi sia a livelli Tutto questo si traduce in una parola per l'Unione europea, e cioè «fragilità». Anche su questo punto il Consiglio europeo dovrebbe discutere seriamente e dovrebbe farlo sulla necessità che non prevalga l'egoismo tra i *partner*, ma si faccia strada l'esigenza che ciascuno rinunci a qualcosa pur

all'ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo. Ma, affinché non siano concetti vuoti, occorrono una presa di posizione più energica del nostro Paese e una consapevolezza certa dei nostri doveri, ma anche dei nostri diritti, che poi sono i diritti di milioni di cittadini che rappresentiamo nelle istituzioni. Per queste ragioni, ci piacerebbe essere più fiduciosi e nutrire speranze, come è giusto che avvenga per tutti noi che siamo chiamati a dare un fattivo contributo alla crescita dell'Unione europea. di insistere sull'interesse dell'Italia di porre al tavolo europeo l'obbligo di resettare e ridiscutere i nostri impegni e la storia della nei decenni. Non siamo euroscettici, anzi ci dichiariamo convintamente europeisti. Ma siamo euroragionatori: pretendiamo, cioè, in nome degli ideali e dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità, di ridiscutere delle nuove politiche finanziarie, di approfondire le visioni sui temi delle politiche industriali e manifatturiere, di valorizzare le produzioni locali, di ridiscutere le politiche bancarie di contrasto delle povertà vecchie e nuove e dell'indigenza diffusa causata dalla lunga e perdurante crisi socioeconomica e finanziaria. In caso contrario, finirebbero per confermarsi le previsioni del professore che lei ha menzionato, insignito quest'anno del premio Carlo Magno. Invece ci aggrappiamo agli auspici di Papa Francesco che, appena qualche giorno fa, ha esortato particolarmente la Germania al dialogo alla capacità di integrazione.

anche le ultime tornate elettorali hanno registrato una battuta d'arresto delle forze populiste. La vittoria di Macron e anche il pessimo risultato nel Regno Unito di Farage, che era stato uno dei principali artefici della Brexit, costituiscono una premessa importante per dare all'Europa quel nuovo slancio di cui ha profondamente bisogno. I risultati elettorali si accompagnano alle previsioni sull'andamento dell'economia europea e al fatto che l'intera area euro sia caratterizzata da una crescita lenta ma costante, con buoni livelli di fiducia che, se accompagnati da politiche mirate, possono portare a un incremento delle spese e degli investimenti. lo credo che tutto questo metta il nostro Paese nelle condizioni di far sentire la propria voce, a partire dal problema dell'immigrazione. Come autonomisti, in questi anni, abbiamo sempre supportato e condiviso il modo con cui questo Governo e quelli che lo hanno preceduto si sono mossi in Europa. Crediamo che un'Europa debole, attraversata da forze centripete, vada a danneggiare soprattutto Paesi come il nostro. Ci vuole l'Europa, ma ci vuole - come ha detto bene, Presidente - un'Europa diversa, più vicina alle istanze dei suoi popoli, sensibile di fronte allo smarrimento per un fenomeno epocale come l'immigrazione, attenta a curare le ferite e le lacerazioni che gli anni duri della crisi economica hanno inferto al nostro tessuto sociale, economico, imprenditoriale. Nonostante alcuni sforzi generosi, nonostante molte dichiarazioni d'intenti, il quadro non è ancora giunto a quella radicale inversione di rotta che tutti auspichiamo. Proprio la scorsa settimana discutevamo in quest'Aula le mozioni sulla Politica agricola comune, evidenziando come a un modello imperniato sulla competitività, sull'innovazione se ne preferisca uno che favorisce le rendite di posizione, la superficie al posto della qualità. È solo un esempio e se ne potrebbero fare altri, ma dà bene la cifra di un'istituzione fredda e impersonale, percepita come troppo distante rispetto ai vissuti e ai bisogni di tanti nostri piccoli e medi imprenditori; un'istituzione che - siamo d'accordo con lei - non si deve accontentare dei decimali di segno più al prodotto interno lordo. Noi crediamo in un'Europa che punta sulla competitività e rimuove ostacoli piccoli e grandi, proprio come è stato fatto con il *roaming*; un'Europa che mette al centro il lavoro attraverso una politica comune di sviluppo industriale e rilancio del settore manifatturiero, che durante gli anni della crisi ha subìto pesanti contraccolpi; un'Europa che si misura con le sfide dell'industria 4.0, dell'Internet delle cose con lo sviluppo della tecnologia 5G, che è in prima linea sui terreni dell'innovazione e della costruzione del mercato unico digitale; un'Europa che ascolti le preoccupazioni dei nostri agricoltori per le ripercussioni che un accordo come il CETA può avere sulle produzioni di grano e sulla qualità dei prodotti che finiscono in tavola; un'Europa che faccia fronte comune nella lotta al terrorismo, anche attraverso il coinvolgimento delle multinazionali del *web*, e non fugga da una gestione collegiale dei flussi migratori. abbiamo molto apprezzato la sua franchezza su questo punto, così come la notizia dell'apertura della procedura d'infrazione a carico di tre Paesi che non rispettano le decisioni comuni. Dall'inizio dell'anno sono giunte via mare nel nostro continente 71.000 persone, di cui 60.000 sbarcate in Italia. Rispetto ai primi mesi dello scorso anno, si è registrata una crescita del 26 per cento ed è aumentato, purtroppo, anche il numero dei minori non accompagnati. Per questo motivo, abbiamo salutato positivamente il provvedimento del ministro Minniti che accelera, finalmente, le procedure di riconoscimento e rimpatrio, ma anche la legge che tutela i minori non accompagnati. insieme, perché danno contezza di un approccio giusto al problema, cioè quello di rispondere in maniera pragmatica alle questioni, senza smarrire i valori di umana solidarietà, ma anche la necessità di dotarci di regole più certe e, soprattutto, di farle rispettare. Siamo d'accordo con lei, signor Presidente del Consiglio, anche sul modo con cui stiamo operando in Libia per affrontare il problema delle partenze. A maggio si sono già visti i primi effetti concreti dell'accordo, in quanto la Guardia costiera libica ha iniziato a intercettare e riportare indietro diverse imbarcazioni di migranti. Bisogna però menzionare anche l'impegno per stabilire accordi bilaterali con i Paesi d'origine per rendere più efficiente la macchina dei rimpatri. È evidente che a questa strategia ancora manca il tassello europeo, che è decisivo e riguarda la stabilizzazione istituzionale della Libia, condizione più che mai necessaria per raggiungere l'obiettivo di chiusura del corridoio che porta fino alle coste italiane. Ma è anche il tassello del diritto d'asilo europeo, perché l'emergenza non può essere scaricata solo sui Paesi d'approdo come il nostro e non può essere sufficiente l'accordo siglato a suo tempo con la Turchia. Il ricollocamento dei profughi, con una distribuzione equa in tutti i Paesi europei, ha interessato, dal 2015 a oggi, solo 20.000 persone, pari a un misero 20 per cento, a fronte di accordi che riguardavano in prima battuta 160.000 persone, successivamente ridotto a 98.000. Adesso si discute se diminuire ancora il numero, portandolo ad appena 33.000. Occorre far sentire la nostra voce, ribadendo che da qui passa molta della credibilità dell'Europa agli occhi del mondo intero. La posizione statunitense sugli accordi di Parigi, i rapporti tra Stati Uniti, Russia e Cina e la minaccia terroristica crescente chiedono all'Europa di giocare un ruolo di primo piano e diventare elemento di stabilizzazione e sicurezza del mondo.

però vivere giorno dopo giorno, attraverso un forte principio di solidarietà e coesione tra gli Stati membri. Per questo, signor Presidente del Consiglio, le chiediamo di continuare con coraggio lungo questa direzione, che il nostro Governo ha ben interpretato anche durante il vertice di Taormina. Sabato scorso, al Sacrario di Castel Dante a Rovereto, abbiamo sepolto i resti di un soldato italiano della Prima guerra mondiale. Il sottosegretario Domenico Rossi e il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Ugo Rossi - come ha fatto il giorno dopo il console generale d'Austria - hanno sottolineato l'importanza di superare i nazionalismi per dare sempre più spazio alla bandiera europea, che è prima di tutto la bandiera della pace; quella bandiera che personalità del calibro di Helmut Kohl hanno saputo riempire di senso e valore, anteponendo l'abbattimento delle frontiere e la politica monetaria comune all'interesse nazionale tedesco e al marco.

Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, le parole pronunciate dal Presidente del Consiglio, anche oggi in quest'Aula, confermano una linea di politica economica improntata alla saggezza e alla responsabilità e rinnovano l'impegno che l'Italia sta portando avanti in sede europea per una crescita più elevata in termini non solo quantitativi, ma anche qualitativi. Con crescita qualitativa intendiamo una crescita basata sulla certezza dell'occupazione, sugli investimenti e sulla produttività, ma soprattutto caratterizzata da una marcata attenzione all'inclusione sociale. La formula più utilizzata, è, per questo, quella di crescita e coesione, quest'ultima intesa come superamento delle fratture e delle distanze sociali che ancora permangono in Europa e che, in Italia, risultano tuttora particolarmente pervicaci. L'unione sociale - si ripete giustamente spesso - si deve accompagnare all'unione economica, monetaria, fiscale, finanziaria. Per la sua creazione sono necessari una revisione e un aggiustamento strutturale del patto di stabilità e delle sue regole: obiettivo da tempo sostenuto dall'Italia insieme alla grande operazione di superamento delle politiche di *austerity* per misure per la crescita e l'occupazione; un superamento da compiere nell'interesse non dell'Italia ma dell'intera Unione. Potremmo dire crescere in modo orizzontale, rendendo ampia la platea di chi partecipa e risente della ripresa. Possiamo affermare che il quadro economico europeo fa registrare un andamento migliore delle previsioni, come certificato recentemente dallo stesso presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi. L'apice della crisi economica è alle spalle, come dimostrano i dati del PIL, e stiamo assistendo, in questo anno, ad una *performance* dell'Europa migliore anche rispetto agli Stati Uniti o al Regno Si stanno raccogliendo dunque risultati positivi, frutto di misure importanti attuate nell'Unione in campo fiscale e monetario. L'Italia ha agganciato questa ripresa, come conferma il Fondo monetario internazionale, che colloca il PIL italiano 1,3 per cento quest'anno, superando le previsioni del più 1,1 per cento prospettate dal Governo stesso. Da mesi gli indicatori della fiducia registrano una crescita, ma in entrambi i casi il margine di fragilità di questa crescita risulta ancora piuttosto forte. Ed è a questo che dobbiamo lavorare, cioè a dare struttura e stabilità alla ripresa. L'Europa infatti cresce ma resta aperto - come accennato prima - il tema della strutturalità della crescita e della coesione sociale. L'Italia cresce ma non abbastanza rispetto agli altri Paesi comunitari.

Per questo la nostra battaglia in sede europea non possiede un asfittico perimetro locale e nazionale, ma assume i contorni e i confini comunitari, riguarda e chiama in causa l'Europa nella sua interezza, la crescita strutturale e stabile di tutti i Paesi che ne fanno parte. Lei stesso, Presidente, ha recentemente ricordato come la richiesta di correzione della matrice necessaria al calcolo del rapporto debito-PIL, per esempio, sia stata il frutto dell'impegno portato avanti dal nostro Paese insieme ad altri Paesi dell'Unione; dunque, tutt'altro che una battaglia solitaria espressione solo di interessi nazionali. Uscire dalla crisi in modo definitivo - dicevamo - è il nostro obiettivo, apprezzando i segnali della ripresa che, per quanto non generino completa soddisfazione, comunque animano la speranza di aver imboccato la strada giusta. Ricordo soltanto i dati evidenziati recentemente dalla Confesercenti nel corso della sua ultima assemblea: in dieci anni sono stati persi 47 miliardi di consumi e il tessuto imprenditoriale italiano è stato decimato, soprattutto a quelle piccole e medie imprese che rappresentano l'ossatura economica del nostro Paese: dal 2007 ad oggi sono state perse 600.000 unità. Sono dati importanti perché senza investimenti per la competitività delle imprese non si realizzano crescita e benessere, non c'è produttività e soprattutto non si crea occupazione. Qui sta il *vulnus* che spiega anche la nostra crescita inferiore rispetto agli altri Paesi europei

che più di tutte le altre tipologie paga chiaramente una esposizione ai temi degli investimenti, dell'innovazione, della ricerca, della produttività e dell'internazionalizzazione.

Penso al nostro impegno nella formulazione del cosiddetto Piano Junker e all'impegno attuale per la sua revisione e il suo ampliamento, non dimenticando altresì azioni concrete che garantiscano una base industriale forte e competitiva, dando piena attuazione all'obiettivo, già fissato dalla Commissione europea, di riportare la quota del PIL europeo prodotto dall'industria manifatturiera almeno al 20 per cento entro il 2020. Sono passi in avanti positivi che necessitano ora di misure capaci di produrre lo scatto definitivo per posizionare la crisi alle spalle, non dimenticando il nostro imprescindibile e doveroso impegno verso il debito pubblico che ancora incide pesantemente sui nostri margini di crescita. In questo senso, la riduzione del carico fiscale sulle imprese rappresenta un traguardo da raggiungere presto, perché garantisce la competitività industriale e favorisce la creazione di posti di lavoro. Non possiamo quindi negare che sarebbe auspicabile la riduzione della pressione fiscale per tutti, ma aggiungo che non si può prescindere da quella alle imprese che - come detto generano occupazione e favoriscono quei presupposti che sono basilari per la coesione sociale, a sua volta basata sulla certezza di lavoro. È questo il meccanismo virtuoso da favorire. A livello europeo continuiamo dunque a insistere per un quadro di politiche fiscali più leggere che diano fiato agli investimenti, che servano loro da ossigeno, tenendo conto che l'ombrello della BCE sul fronte monetario (in particolare la sua seconda *tranche*) andrà progressivamente a ridursi e l'Europa dovrà prepararsi ai possibili contraccolpi dando una risposta. Avviandomi alle conclusioni, signor tema altrettanto centrale è quello rappresentato dalla sfida della banda larga: per l'Italia, così come per l'Europa, è essenziale la sfida della digitalizzazione. La strategia per il mercato unico digitale deve essere realizzata per migliorare l'accesso ai beni e servizi digitali in tutta Europa per i consumatori e le imprese e per massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale. gli ultimi mesi sono stati delicatissimi per l'Europa - come da lei ricordato, un anno fa - perché il *referendum* britannico perché la Brexit poteva innescare un sistema distorsivo, alimentando quelle forze populiste che minano la credibilità delle istituzioni, diffondendo la falsa percezione fra i cittadini che sia l'Europa il nemico, un'Europa ridotta a tecnocrazia e raccontata esclusivamente come potere di ricatto burocratico. È una falsità, perché la verità politica è esattamente opposta: fuori di essa non esiste futuro economico per i nostri Paesi. Certo non sfugge - e il nostro Paese è impegnato su questo fronte, come ho ricordato all'inizio del mio intervento - la necessità di un cambiamento perché l'Unione diventi sociale e politica, completando un processo di unificazione frutto di un lungo e virtuoso cammino, di cui recentemente, a marzo, abbiamo celebrato i sessant'anni, perché - come diceva lei, signor Presidente - non ha suonato una campana a morto, ma c'è stata una robustissima sveglia.

il voto che avrebbe potuto mettere in crisi l'Europa unita, cioè quello francese, è stato fortunatamente superato oltre ogni previsione. Le forze populiste sono state di fatto ridotte a una minoranza ininfluente e ciò grazie a Macron che ha sfidato i populisti e le vecchie forze politiche proprio in nome dell'Europa, senza reticenze.

che oggi il vero discrimine fra le forze politiche è tra una visione aperta e europeista della società - da un alto - e una prospettiva chiusa e nazionalista, dall'altro. E io credo che, se Angela Merkel riconfermerà il suo successo - in ogni caso la Germania non ha grandi problemi - Francia e Germania potranno dare un nuovo impulso all'unità europea, con politiche che guardano alla crescita senza però tralasciare la necessità di mettere in sicurezza i conti pubblici. E l'Italia può e deve essere nella partita, ma dovrà dimostrare di essere capace di proseguire il cammino delle riforme, come lei, presidente Gentiloni Silveri, sta facendo, facendo, nonostante la bocciatura della riforma costituzionale che - non lo dimentichiamo - avrebbe potuto assicurare all'Italia, come alla Francia, un sistema politico più stabile e forte. Lasciatemi dire, colleghi, che non passa giorno in cui io non mi capaciti di un errore così grande che l'Italia ha commesso nel bocciare la riforma.

come l'approvazione della legge sulla concorrenza e della legge di stabilità, con forti provvedimenti a favore delle imprese e dell'occupazione giovanile, a cominciare dal taglio del cuneo fiscale, che anche lei ha annunciato. Resta, però, presidente Gentiloni Silveri, la rilevante questione dell'immigrazione che pesa troppo sulle nostre spalle e viene strumentalizzata ogni giorno da un'opposizione che dimentica di aver governato da decenni. Su questo piano l'Europa non può continuare a girarsi dall'altra parte ma deve assumersi le sue responsabilità. L'Italia non ce la può fare da sola. Come abbiamo detto tante volte, rischia di fornire così un argomento troppo forte alle forze populiste e di destra, che speculano senza ritegno su una questione delicata come questa.

Da questo punto di vista, la nuova Europa, anche con Macron, ci può dare un aiuto di stile e soluzioni.

c'era). Vorrei ricordare che un anno fa, e anche prima, c'erano non toni concilianti, bensì un vero e proprio terrorismo e bullismo da parte della Commissione europea (organo notoriamente democraticamente eletto),

ci sarebbe stata una svalutazione della sterlina; la borsa della Gran Bretagna sarebbe andata a picco e i titoli Gilt non sarebbero stati più piazzati sul mercato. Ne aveste azzeccata una, anche per sbaglio: neanche una. Neanche tirando a indovinare uno può sbagliarle tutte. Questo vuol dire che, intenzionalmente, si fa propaganda.

tutte le volte che si crea questo tipo di categoria si sta facendo propaganda. Quindi, a proposito di propaganda, la Commissione europea e il Parlamento europeo nel 2013 hanno approvato un documento, reperibile sulla rete, dove è scritto che sono stanziati (e sono stati stanziati) due milioni per fare un monitoraggio di tutti i *social network* volto a individuare i *troll* antieuropeisti ed euroscettici e bloccare tutti questi tipi di discussione, arruolando a propria volta pattuglie di *troll* per fare questo. Nel 2016, il Parlamento europeo ha approvato un'altra risoluzione nella quale dice che bisogna continuare questo tipo di attività di controllo, monitoraggio e repressione della propaganda anti UE da parte di terzi. In altre parole, non esiste un dibattito equo sull'Unione europea, esiste la propaganda e la lotta contro la propaganda avversa.

In letteratura scientifica ci sono centinaia e centinaia di pubblicazioni sulle più importanti riviste economiche del mondo che hanno smantellato, dall'inizio alla fine, tutti i dogmi e la propaganda sull'euro e sull'Unione europea. Le faccio un esempio giusto per chiarire: lei ha lodato

parola "superpotenza" evoca il concetto di suprematismo, di supremazia su qualcun altro, e quindi di competizione tra individui sempre più grossi. E chi sono i nostri competitori? Lei non lo ha detto, ma lo dicono tutti gli altri propagandisti pro UE che parlano di competitori, come la Cina da una parte e gli Stati Uniti e il blocco NAFTA dall'altro. Bene, visto che gli Stati Uniti non sarebbero contenti dell'introduzione dell'euro, le voglio ricordare una pubblicazione scientifica che è apparsa nel 2006 sulla rivista «American Economic Review» che raccoglie le opinioni dei più grandi economisti americani in un arco di tempo piccolo, dal 1989 al 2002. La stragrande maggioranza di questi economisti ha dichiarato che l'euro era una cosa buona, non una cosa cattiva. L'euro, è vero, è apparso ufficialmente nel 1997 (anche se poi l'abbiamo visto in tasca solo nel 2002), perché quell'anno siamo stati ancorati stabilmente, per obbligo, alla parità con quello che si chiamava Ecu a 1936,27 lire. Quindi abbiamo avuto un lungo periodo nel quale vigeva tale obbligo e agli Stati Uniti, nostri concorrenti osteggiatori dell'euro, questo andava bene:

Questo è un giudizio di merito e morale. Non esiste un europeismo riluttante, esistono libere persone con un libero pensiero, che magari non sono allineate con il pensiero pro UE che non vuol dire pro Europa. L'Europa, infatti, è un'unità fisica e tutti noi, nati in questo continente, siamo europei e basta. Non è un concetto legato alla nazionalità. Semmai dobbiamo distinguere euro, Unione monetaria, Unione europea ed Europa. Non facciamo confusione. Le dico questo perché nel momento in cui si fa questo non si fa un servizio ai cittadini, perché è propaganda. Ma andiamo avanti, perché è giusto andare avanti. Lei ha detto che si pensava che l'Unione europea fosse il problema. ha aggiunto che ora, invece, è cambiato tutto. Le chiedo: cosa è cambiato? Le carte che erano sul tavolo un anno fa sono le stesse che ci sono adesso: non è cambiato assolutamente niente.

invece di favorire l'armonia intra-UE e una pace globale, è molto più probabile che il passaggio all'Unione monetaria e la conseguente integrazione politica conducano ad un aumento dei conflitti intra-UE. Ebbene, è successo: i conflitti intra-UE sono costanti, sono naturalmente conflitti relativi al commercio interno e alla moneta unica che, alla fine,

M5S)*. Se vogliamo fare un dibattito sullo stato della UE e dell'unione monetaria, almeno facciamolo equo: diamo a tutti quanti la possibilità di conoscere le cose. Non pretendo che uno vada a leggersi gli scritti e le pubblicazioni scientifiche - ci sono un sacco di riviste perché si pubblica tantissimo nel mondo

siamo stati quelli che hanno comprato le merci tedesche indebitandoci perché, non potendo produrre nuovo debito, abbiamo dovuto agire sui salari facendo deflazione e abbiamo dovuto creare debito. Quindi anche in questo caso, quando si viene a dire che è importante che l'investitore estero investa in Italia, è un'altra frase fatta. Cosa vuol dire che l'investitore estero investe? Che ti sta prestando soldi suoi.

Senatore Martelli, prego, riprenda il suo intervento. Grazie, Presidente, chiedo scusa per essere stato interrotto. Dicevamo: quando un'azienda cinese compra un pezzo di un'azienda italiana, vuole un *payout* in termini di pagamento del dividendo, quindi, di fatto, c'è un drenaggio di capitali da noi verso la Cina.

la conquista di spazio geopolitico da parte dell'Unione europea, vorrei fare un'osservazione nel merito. L'Unione europea non ha acquisito uno spazio geopolitico. Addirittura, si è dimostrata incapace di dirimere questioni interne come, per esempio, il concetto di migrazione, che lei, presidente Gentiloni due esempi che ci fanno capire come l'Unione europea non sia altro che un randello finanziario e l'euro non è una moneta, ma uno strumento di controllo e vado ad argomentare. Con la Grecia, che ha l'euro,

allora, invece di continuare ad affidarsi al medico che ti ha fatto ammalare sperando che ti guarisca, si molli quel medico e si provi a ricominciare da zero. *(Applausi Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, abbiamo apprezzato la pacatezza e l'attinenza al tema delle sue comunicazioni, cosa a cui non eravamo sempre usi negli ultimi anni. Abbiamo apprezzato nel contenuto alcuni aspetti delle sue comunicazioni, in particolare l'accenno alla necessità di tenere un atteggiamento pragmatico sulla Brexit, né *hard* né *soft* Brexit, ma una una Brexit che sia sensata e che, in particolare, difenda gli interessi degli italiani che si trovano nel Regno Unito e, in generale, i rapporti fra le imprese e le persone italiane con il Regno Unito. un atteggiamento molto più apprezzabile rispetto ad alcuni alti esponenti dell'Unione europea, che hanno auspicato un atteggiamento di vendetta nei confronti del Regno Unito. La vendetta è cosa poco razionale in generale, ma tanto più è in politica e tanto più nella politica internazionale, per un legittimo atto che i cittadini del Regno Unito a maggioranza hanno deciso di intraprendere. Noi non soltanto apprezziamo, ma sosteniamo e stiamo sostenendo

parte importante della Giunta, sta sostenendo attivamente, fattivamente e concretamente questo tentativo che noi riteniamo meriti di avere successo, portando a Milano queste importanti agenzie europee. Speriamo

senza consultare a quanto pare nessuno, svantaggiando enormemente le banche italiane e lo Stato italiano, senza che ce ne fosse una ragione nell'economia reale. Noi sosteniamo chiunque sieda fra i banchi del Governo, quando fa gli interessi del nostro Paese. Abbiamo apprezzato anche il ricordo di Helmut Kohl. Dopo l'intervento del Presidente del Consiglio ci sono stati altri che hanno citato la figura di Helmut Kohl, una figura estremamente importante: senza di lui, l'Europa sarebbe stata diversa e la storia dell'Europa sarebbe stata diversa. Sono contento del fatto che oggi, a trent'anni dal vertice della carriera politica di Kohl e a pochi giorni dalla sua dipartita, ci sia questo ampio apprezzamento nei confronti Ricordo che a suo tempo, quando era candidato (a volte vincente e a volte no) del centrodestra tedesco, cioè dei cristianodemocratici tedeschi, contrapposto alla sinistra dei socialdemocratici,

intellettualmente inferiore rispetto ai fulgidi luminari che c'erano nella sinistra. Questo è un vizio che scontiamo per l'Italia come per la Germania: sono sempre dei geni quelli che stanno a sinistra. Però Helmut Kohl, sia pure trent'anni dopo, vedo che riscuote

difenderanno con il loro voto un provvedimento che prevede, per chi fosse anche solo sospettato o indiziato di alcuni dei fatti che poi coinvolsero Kohl a proposito del finanziamento del suo partito,

in anni di carcere, gli venga sequestrato il patrimonio e tolto il sostentamento per la vecchiaia. Detto questo, ricordiamo che quando Kohl ha avuto un ruolo attivo, fin tanto che l'ha avuto, nel nel determinare la fisionomia dell'Unione europea, ha lavorato perché essa fosse realmente ispirata ai criteri di solidarietà e coesione,

il presidente Trump. A proposito degli accordi di Parigi, credo che l'uscita degli Stati Uniti dovrebbe essere lo spunto se non per rinegoziarli, perlomeno per farsi qualche domanda: come mai negli accordi di Parigi la Germania, che ha il 36 per cento di abitanti in più dell'Italia, può avere emissioni del 98 per cento superiori a quelle dell'Italia? Se l'è mai chiesto qualcuno? È stato mai chiesto in sede europea come mai?

per dare un'occhiata a questi meccanismi? È logico che negli accordi di Parigi la Cina e l'India, che già oggi hanno emissioni altissime (la Cina il doppio degli Stati Uniti e cioè 26 volte l'Italia), possano continuare a farle crescere fino al 2030? Bellissima cosa l'atto di fede a favore dell'accordo di Parigi, ma oltre a professare atti di fede, oltre a farsi applaudire nelle sedi internazionali, chi rappresenta l'Italia dovrebbe difendere gli interessi dell'Italia, esattamente come il celebrato Helmut Kohl difendeva gli interessi della Germania in un'Europa solidale, quella dei suoi tempi.

l'Italia vuole fare il primo della classe su una serie di punti? Qualche settimana fa è stata approvata la legge sui minori - o meglio sugli autodichiarati minori - stranieri non accompagnati, esponenti della maggioranza e del Partito Democratico hanno vantato che si tratta di una legge all'avanguardia in Europa, quando è una legge molto, ma molto più lassista di qualunque altro Paese europeo. E poi diciamo che abbiamo bisogno di una politica europea comune. Andiamo a prendere - unico Paese al mondo e nella storia le persone che vogliono venire dall'Africa in Italia a ridosso della costa africana, ma poi pretendiamo che gli ungheresi si prendano la loro quota. Questo non va tanto bene. Per non parlare, poi, della legge chiamata *ius soli*, che in realtà è molto più ampia dello *ius soli*,

Signor Presidente, signori del Governo, colleghi senatori, questo Consiglio europeo avviene in un momento molto particolare, in cui si colgono i segni degli effetti della nuova presidenza americana, le conseguenze della Brexit, della svolta leaderistica in Turchia, delle elezioni francesi, della guerra diplomatica in corso nel Golfo tra i sunniti, ma anche in relazione alla componente sciita. Segni che ci chiamano, come italiani ed europei, ad essere all'altezza di sfide a cui bisogna rispondere con strumenti nuovi, ancorandoci a certezze antiche. La certezza antica è che non c'è futuro fuori dall'Unione europea e contro l'Unione europea; che l'Europa si cambia partendo da questa Europa; che l'aggressività di antichi alleati (penso agli Stati Uniti e ai rischi di un loro ripiegamento protezionistico e nazionalistico sempre più evidente) e nuovi *competitor* richiede una fase nuova del processo di integrazione europea, che passa anche attraverso l'agenda del prossimo Consiglio europeo. Certo, non possiamo attenderci decisioni rivoluzionarie, ma il mutato clima nei confronti dell'ineluttabilità del tramonto dell'Unione europea chiama i Governi europei e le istituzioni dell'Unione a un impegno più forte per dare attuazione alla dichiarazione di Malta sulle migrazioni, per arrivare a una normativa comune sul diritto di asilo, per dare corpo a un piano per l'Africa che sani le antiche ferite del nostro colonialismo e contenga la vocazione espansionistica soprattutto di India e Cina sul continente africano, incoraggiando la crescita dell'Africa. Anche la crescita dell'Europa dipende sempre più dal rafforzamento del processo di integrazione politica, che, fin dal prossimo Consiglio europeo, vuol dire completamento dell'unione monetaria e bancaria, avvio di una vera unità fiscale, rafforzamento del bilancio dell'Unione europea, perché non esiste un rafforzamento politico dell'Unione europea senza più risorse per accompagnare la crescita con adeguati investimenti, per un debito pubblico europeo solidale e condiviso. In questo quadro, l'uno per cento del PIL europeo a favore del bilancio dell'Unione europea non consente di realizzare le politiche che pure auspichiamo. Di questa ripresa di iniziativa politica hanno bisogno non solo gli Stati e i popoli del vecchio continente, ma anche il mondo intero. Non può non esistere una Europa politica forte per contrastare rigurgito di guerra fredda cui stiamo assistendo, in cui la guerra digitale si affianca a quella tradizionale, per cercare nuove egemonie e in cui la imprevedibile e subdola strategia terroristica dei gruppi islamici più estremisti sta seminando morte in Europa e in Occidente. In questo quadro, il rafforzamento del sistema di difesa e di relazioni esterne dell'Unione europea richiede decisioni più determinate, più veloci di quanto fin qui è stato. Anche da questo Consiglio europeo ci aspettiamo indicazioni chiare sugli obiettivi che ci si vuole dare per un nuovo sistema di difesa europeo, che riprenda il sogno spezzato sogno spezzato nel 1954 con la fine della CED e che getti le basi di una svolta verso quell'unione politica che resta il traguardo finale del processo di integrazione europea. Solo da una svolta nella definizione degli obiettivi, nella convinzione nel perseguirli, soprattutto da parte di Germania, Francia, e Italia che con i loro 200 milioni di abitanti sono il cuore dell'Europa di oggi, dopo la Brexit, possiamo sperare di avere la forza di porre in essere quelle politiche di crescita, senza le quali l'Europa non solo rischia di non essere più la prima economia del mondo, ma rischia anche di perdere quell'insostituibile primato che ha nel saper coniugare livelli di benessere, libertà politica e protezione sociale. C'è grande spazio ancora per rafforzare il mercato interno, per superare le barriere non tariffarie tra i nostri sistemi economici ed eliminare i piccoli e grandi *dumping*, che alterano la concorrenza all'interno dell'Unione europea e impediscono o alterano un corretto accesso al mercato. però essenziale per l'Unione europea utilizzare il proprio peso politico ed economico per aprire gli altri mercati, rimettere al centro l'impegno a favore del multilateralismo, utilizzando anche gli accordi di libero scambio per favorire pace e sviluppo, dimostrando che la dottrina Trump è negativa per gli Stati Uniti e per il mondo e che il protezionismo, per l'Europa e soprattutto per un'Italia povera di materie prime, è il più grande ostacolo alla crescita e quindi all'occupazione e alla riduzione del debito pubblico, che la crisi finanziaria ci ha lasciato in eredità. Signor Presidente, colleghi senatori, i risultati elettorali di Paesi europei molto importanti ci hanno dato la chiara indicazione della strada da percorrere. Speriamo di non essere l'eccezione che conferma la regola, ma la strada è chiara. Il processo di integrazione non deve fermarsi e l'Unione europea va completata, il populismo si sconfigge raccontando la verità ai cittadini ed esaltandone il senso di responsabilità. La storia dell'Europa è una storia di *stop and go*. È stato così dopo la sconfitta della Comunità europea di difesa (CED), con la contrapposizione franco-inglese e con la bocciatura del progetto di Costituzione. Dopo sono però venuti i Trattati di Roma, l'Atto unico e il Trattato di Lisbona. È tempo di pensare al domani, senza dimenticare le emergenze quotidiane e questo domani occorre costruirlo oggi, ponendoci anche il problema di come rafforzare ulteriormente la dimensione democratica dell'Unione europea. Occorre arrivare alle elezioni del 2019 con un'idea guida forte su come meglio equilibrare il potere di iniziativa, che di diritto spetta alla Commissione, l'organo comunitario per eccellenza, ma che di fatto oggi è nelle mani del Consiglio, vale a dire dei Governi nazionali, quegli stessi Governi che spesso hanno trovato una via d'uscita più semplice dai problemi, additando l'Europa come causa dei problemi stessi, piuttosto che come loro soluzione. In questi anni l'Europa ha rischiato di essere travolta dall'asfissia inconcludente della dimensione intergovernativa. Se c'è qualcosa che dalla lezione dei Padri fondatori dobbiamo recuperare davvero

se ampliamo i poteri di iniziativa del Parlamento e restituiamo alla Commissione un vero ruolo di governo. Rafforzare la dimensione democratica vuol dire anche coinvolgere sempre di più e meglio l'opinione pubblica nella narrazione di questo tempo, anche con consultazioni su problemi specifici, ad esempio in occasione delle prossime elezioni europee, come peraltro già è avvenuto in passato.

difenda l'accordo di Parigi sul clima e apra un confronto a tutto campo con gli Stati Uniti su questo tema e su quello del commercio mondiale, pensi alla migrazione dall'Africa non come ad una pertinenza biblica, ma come la cartina di tornasole del bisogno di una nuova logica distributiva delle risorse e delle ricchezze del mondo. Essere alla testa di questo processo epocale è il dovere di un grande Paese, che sa alzare lo sguardo oltre le proprie meschinità. Siamo sicuri che voi, signori del Governo, e lei, signor Presidente del Consiglio, ne siate più che consapevoli e confidiamo che l'approccio assai positivo assunto in questi mesi sulle questioni europee e internazionali, non solo darà centralità al ruolo dell'Italia, ma rafforzerà quella flebile speranza, che abbiamo visto rinascere in Europa e che ci fa ritenere che il tempo del tramonto dell'Unione europea e dei tuoi Stati non sia ancora all'ordine del giorno.

testi sono in distribuzione. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

occorre evitare una permanente»;

alla risoluzione n. 5, non condivido praticamente nulla di quanto ha detto il senatore Martelli, ma condivido molto di quanto è indicato nella risoluzione, perché sono tante azioni che il Governo ha in corso quindi, se i proponenti accettano le riformulazioni del Governo, il parere è favorevole.

Per quanto riguarda il dispositivo, dato che si tratta di azioni su cui il Governo sta lavorando, propongo riformulazioni che rendono più attuali gli impegni proposti dai proponenti. riformulato come segue: «a continuare nell'impegno volto a superare l'attuale sistema di Dublino e a rivedere in particolare il principio del "Paese di primo approdo", valutando anche la possibilità di permettere

Signor Presidente, condivido quanto è stato detto nei punti principali della discussione di questa mattina. Vorrei però fare delle alcuni aspetti, innanzitutto sulla Brexit. A quasi un mese dall'ultimo intervento del presidente Gentiloni in Aula, in occasione del quale chiesi di fare chiarezza sui costi della Brexit, torno, dopo le note polemiche proprio su questo tema, a chiederle di far sì che il presidente Gentiloni in prima persona si faccia portavoce di questa necessità che è propria di tutti i 27 Stati membri. È necessario fare il punto su quanto la Brexit costerà alla nostra economia, all'economia dell'Unione, come è necessario sapere quali risposte dare ai nostri connazionali che nel Regno Unito vivono e lavorano e che, ad oggi, ancora non hanno chiaro quale sarà la disciplina applicata al loro inalienabile diritto di libera circolazione. I negoziati, iniziati qualche giorno, fa, non devono essere occasione per esprimere risentimento, ma occasione di onesto confronto sul tema, tenendo presente che la tenuta del nostro sistema economico deriva direttamente dall'approccio che l'Unione europea deciderà di tenere con il Regno Unito. il Regno Unito. La migrazione è un altro tema all'ordine del giorno del Consiglio europeo e sarà necessario fare una valutazione per attuare le misure da adottare per arginare i flussi migratori lungo la rotta del Mediterraneo centrale. A fronte degli ultimi dati forniti dall'Organizzazione internazionale delle migrazioni, risulta ad oggi che nel Mediterraneo nel 2017 ci sono stati 2.000 morti, oltre 81.000 arrivi di migranti, di cui l'85 per diretti in Italia. Mi pare evidente che l'Italia debba impegnarsi affinché cambi radicalmente il modo di affrontare l'emergenza. La volontà dell'Unione è quella di non rivedere gli accordi di Dublino, rideterminando il numero di richiedenti asilo destinati ad ogni singolo Paese, ma l'Italia non può reggere da sola il peso dell'85 per cento di questa emergenza. Aggiungo che più che analizzare le politiche di intervento nel Mediterraneo centrale, il vero grande tema da affrontare è quello della cooperazione e dello sviluppo del continente africano. Solo una forte *partnership* economica e sociale tra Europa e Africa, a guida italiana, e non le elemosine che da troppo tempo siamo abituati ad elargire, può assicurare il vero controllo del fenomeno migratorio. È inutile continuare a valutare interventi limitati ad un ripescaggio quotidiano da parte delle nostre Forze dell'ordine e della nostra Guardia costiera, alle quali però va tutta la nostra gratitudine per il loro impegno, che ci consente di affrontare a testa alta il tema nelle sedi europee. L'Italia deve ottenere, tramite il nostro Presidente del Consiglio, un vero impegno dell'Europa nei Paesi dai quali i barconi partono, per assicurare condizioni di vita dignitose alle popolazioni che, anche a causa di talune politiche estere, scappano dalla propria casa, dai propri valori, dai propri affetti e cercano di raggiungere un Paese che non è in grado di accogliere, in sei mesi, quasi 57.000 migranti. Questo, peraltro, non è un indirizzo di politica di destra

Non possiamo consentire che si muoia al largo delle nostre coste, come non possiamo sostenere un fenomeno che non è assolutamente solo italiano, ma di cui l'Italia sopporta il maggior peso. Noi tutti guardiamo con inquietudine ai preoccupanti eventi terroristici che stanno sconvolgendo il continente. Non è questo il luogo per dibattere demagogicamente sulle cause di questa *escalation*, però l'Italia avrà l'occasione di essere faro guida nella prevenzione del terrorismo e degli attacchi: la grandissima esperienza che il nostro Paese ha potuto, suo malgrado, fare negli anni bui della nostra storia repubblicana in tema di prevenzione e sicurezza dei cittadini e delle istituzioni deve essere messa a disposizione dei nostri alleati. alleati. Come per molti degli altri settori, occorre molta più Europa. Siamo rimasti fermi all'Interpol, lasciando che i servizi di sicurezza nazionale non si parlassero. Se non capiamo che maggiore integrazione significa più risultati, l'esito sarà sempre deludente. Da ultimo, in occasione del semestre europeo 2017, è necessario continuare a portare avanti una lotta che consenta all'Italia di attuare vere politiche mirate all'occupazione, alla crescita e alla competitività, *in primis* con riferimento alle nostre eccellenze, alle nostre esportazioni, al marchio *made in Italy* che l'economia del dell'Europa teme. È vero che il nostro Paese ha accumulato un grandissimo ritardo, ad esempio nella digitalizzazione delle imprese. Confindustria digitale calcola una perdita dal 2000 al 2015 di 200 miliardi di euro a causa di questo. Per questo motivo l'Unione deve consentire all'Italia, in tempi e con modalità che non sviliscano la nostra economia, di adeguarsi agli *standard*. Lo stiamo facendo con il piano Calenda, ma abbiamo bisogno di più sostegno dall'Europa perché ulteriore sostegno all'Italia è ulteriore sostegno a tutta l'Unione. È necessario infine... PRESIDENTE. Concluda. Grazie, Presidente, verrebbe da parlare di vuoto assoluto, che è un po' anche quanto ci ha ricordato prima in maniera molto laconica il presidente Gentiloni Silveri: da solo, senza alcun Ministro attorno

un guscio di noce messo in acqua aspettando che vada a schiantarsi contro gli scogli, con anche da parte della maggioranza qualcuno che fa il tifo perché gli scogli si avvicinino il più velocemente possibile. Noi non giochiamo al tanto peggio tanto meglio. Vorremmo invece, almeno in questo ultimo scampolo di legislatura (visto che avete deciso di trascinarla ancora per qualche mese), che il Governo facesse la propria parte, difendendo gli interessi dei cittadini italiani

altrimenti il Paese non può ripartire. Quella flessibilità è arrivata, i fondi sono stati messi a disposizione, ma non sfuggirà nessuno cosa sta succedendo, basta prendere un quotidiano e leggerlo: sisma, caos e ritardi. Cantone e l'antimafia indagano sui subappalti per casette e macerie. Questo è un quotidiano di oggi, signor Presidente.

il fatto che devono essere almeno esentati dal pagamento delle tasse di successione i poveri disgraziati che sono rimasti sotto il terremoto. Questa è la serietà del Governo. Questa è la serietà che il Governo ha messo nella ricostruzione delle aree terremotate. terremotate. Ma se questa è la serietà che il Governo ha messo su una questione così importante, non è difficile comprendere quanto il Governo non sia credibile su altre tematiche nel momento in cui si rivolge all'Europa chiedendo flessibilità, impegnandosi sul fronte economico piuttosto che su quello della ripresa sociale e finanziaria. Presidente Gentiloni Silveri, il problema è che non siete credibili non siete credibili perché è in ciò che fate, ovvero in ciò che non fate, che dimostrate di non essere credibili. Proprio ieri, non più tardi di qualche ora fa, in quest'Aula andava in onda lo psicodramma di maggioranza, con parte della maggioranza che votava contro lo stesso Governo per le mozioni riguardanti lo scandalo Consip, e parte della maggioranza, il PD, che chiedeva una verifica.

Se non sgombrare il campo velocemente da questi fantasmi, il problema non è che andrete a fondo voi, ma che porterete a fondo tutto il Paese insieme a voi. Cominciate a cacciare Errani e a cacciare Lotti e iniziamo a dare un segno di discontinuità rispetto a una gestione che sta facendo solo danni gestione che sta facendo solo danni al Paese. La serietà la si dimostra pagando i fornitori e non essendo l'ultimo Paese in Europa per il ritardo dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione.

La nostra economia, rispetto a quella di un altro Paese come la Spagna, che è entrata in crisi tanto quanto noi all'inizio degli anni 2000, sta arrancando, mentre in quel Paese ormai ha ripreso il volo. Qual è la differenza? È nelle scelte politiche di base.

All'ordine del giorno del Consiglio europeo vi sono questi temi. Il primo è ancora una volta la migrazione. Ogni volta che c'è un Consiglio europeo il primo tema è la migrazione. E quali sono le risposte? Ogni volta, il nulla. può anche continuare a dire che l'Europa ha ripreso con vigore e che l'antieuropeismo è stato sconfitto. L'antieuropeismo non è un fenomeno stagionale come le foglie che crescono e cadono. Il problema è l'Europa che non riesce a risolvere i problemi e i cittadini che non hanno fiducia in un meccanismo fatto solo di burocrazia e di grandi interessi, non di tutela dei più deboli e dei più fragili. Oggi abbiamo avuto, ancora una volta di più, la conferma del fatto che l'Europa si basa sulla finanza, mentre noi, nel primo articolo della Costituzione, abbiamo scritto che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Voi oggi state portando l'Italia a rinunciare alle proprie basi fondanti, al riconoscimento del lavoro come la vera fonte di dignità per le persone sottoponendo invece l'Italia a vincoli finanziari.

Ma qual è la serietà del Governo in merito alla sicurezza quando, con il riordino delle carriere, avete creato uno scompiglio nelle Forze dell'ordine e, ancor peggio, un salasso nei loro confronti? Quali motivazioni date ai nostri agenti nelle strade, cui chiediamo, e chiedete, tutti i giorni di mettere a disposizione la loro competenza, la loro professionalità e di mettere a rischio anche la loro vita per difendere i cittadini, quando non consentite loro neanche di programmare il *budget* della propria famiglia perché li salassate? Questa è la serietà con cui poi governate il Paese e con la quale vi rivolgete all'Europa. Ma dove credete di andare? Ribadisco: fosse solo il problema della vostra maggioranza che va a picco! Ma il problema è che portate a picco l'intero Paese con questo vostro modo di concepire la politica.

allo scemo della combriccola quando viene accolto dagli altri. Questa, purtroppo, è l'immagine che oggi deriva quando vediamo il nostro Paese rappresentato in Europa. Avremmo voluto vedere discusse qui dentro le mozioni riguardanti l'agricoltura e la filiera del riso, ma per l'ennesima volta sono state posticipate. Ancora una volta state danneggiando il nostro Paese non difendendo il lavoro di chi, a partire dall'agricoltura, paga le tasse, mettendoci sudore e fatica, chiedendo semplicemente di essere riconosciuto e rispettato nella propria capacità di lavorare e di creare ricchezza. A voi, invece, questo non interessa. Va bene che l'Unione europea non metta i dazi e consenta le importazioni di riso dalla Birmania mandando a fondo l'intero comparto e se poi chiudono le imprese e restano a casa restano a casa i nostri lavoratori chi se ne importa, tanto per voi è importante che venga qualche finanziatore dall'estero, meglio se poi collegato anche a Renzi e ai suoi amici delle banche, ad acquistare in saldo le imprese italiane. Questo non è quello che si chiama un Governo serio.

Prima ce ne liberiamo, prima si torna al voto e prima potremo tornare nell'Unione europea a dire che gli interessi dei cittadini italiani, dei cittadini del nostro Paese, vengono prima di quelli degli altri.

e quindi, a maggior ragione, voglio ribadire oggi la condivisione nei confronti degli orientamenti che ha esposto. Vorrei prendere le mosse da un'affermazione del suo intervento: intervento: il Presidente ha definito l'Europa "un progetto centrale del nostro futuro". Trovo particolarmente stimolante questa osservazione, perché sono convinto che l'identità dell'Europa non appartenga soltanto al suo passato, ma sia iscritta nel suo futuro. C'è un passaggio molto Europa» di Edgar Morin e di Mauro Ceruti, che è stato nostro collega senatore, nel quale i due studiosi sostengono che l'Europa non sia più un bruco, nel senso che è uscita dalla propria crisalide, ma non è ancora una libellula. Credo che questa immagine ben dica delle sfide e degli appuntamenti che ci attendono. Dicevo una grande storia, perché l'Europa affonda le sue radici persino nella tradizione mitologica, nel mito di Cadmo e Armonia, ed è al centro, è il luogo d'origine dei processi di mondializzazione e di occidentalizzazione. Possiamo parlare di un'Europa che è ovunque - l'eurasia, le euro-americhe,

energetiche e per quanto attiene alla sua vocazione, che, non può essere disconosciuta o negletta, di grande potenza. Ebbene, quali sono le premesse perché l'Europa possa affrontare le sfide sull'arco complesso dei problemi che il Presidente, con grande nettezza e credo onestà intellettuale, ci ha presentato? Innanzi tutto l'Europa ha davanti a sé una sfida, la necessità che essa diventi un plebiscito quotidiano, per parafrasare una definizione che in passato è stata data della democrazia,

rassicuranti anche se mi permetterò qualche chiosa) deve essere il continente che abroga la dimensione del rifiuto e che è in grado di proporre oggi un *new* *deal* europeo. europeo. L'Europa che non è una provincia, è l'Europa che affronta la grande sfida del nostro tempo, cioè la sfida della globalizzazione.

l'Europa che rilancia le prospettive della propria economia sociale di mercato. È un'Europa che rilegge ‑ questa è una sfida che compete a tutti noi ‑ il grande tema della globalizzazione, che certamente abbiamo interpretato, in un passato anche recente, esclusivamente in termini di eccellenza, di merito, di flessibilità, e che oggi invece credo ci ponga la sfida di un'Europa come grande Stato innovatore, come grande Stato che persegue di investimenti, che assume l'ambizione della crescita, che pone rimedio al mondo globalizzato delle diseguaglianze, delle fragilità, delle difficoltà che investono milioni di cittadini e di persone. Quando giustamente si parla - ed è un obiettivo degno di essere perseguito - di unione economica e monetaria, non basta. Bisogna definire quale declinazione si dà, appunto, a questi obiettivi. Io credo che centrale debba essere l'Europa della crescita, l'Europa del lavoro, l'Europa del riscatto della dignità dei propri cittadini. Giustamente, il presidente Gentiloni Silveri ha richiamato un panorama internazionale profondamente mutato e che problematizza uno degli assi fondamentali della politica estera europea: l'asse della politica transatlantica, perché le scelte di Trump, le scelte di un protezionismo di ritorno alla vecchia dottrina di Monroe, interrogano l'Europa e credo che la risposta sia più Europa, più integrazione, più capacità dell'Europa di porsi a riferimento della possibile soluzione dei grandi, epocali problemi del nostro tempo. Sotto questo profilo mi pare che la vittoria di Emmanuel Macron in Francia costituisca per noi un fattore di rassicurazione, perché Macron ha vinto sulla base non di uno *slogan,* ma di un progetto, che è il progetto di più Europa, non di meno Europa. Così pure il deludente risultato - deludente a dir poco rispetto alle sue originarie ambizioni - di Theresa May ci pone, anche in questo caso, di fronte alla sfida della Brexit, che è la sfida del mantenimento degli impegni finanziari, della tutela e della promozione dei diritti dei cittadini europei, e dunque italiani, residenti in Gran Bretagna. È la sfida dell'armonizzazione del diritto europeo e del diritto della e del diritto della Gran Bretagna; la sfida del mercato unico, dei confini tra l'Ulster, l'Irlanda. Ebbene, il tema della Brexit ci pone oggi di fronte a una inedita possibilità, alla luce del fallimento dei propositi di *hard* Brexit, e cioè la possibilità di definire una sorta di divorzio amicale nel mantenimento degli impegni assunti anziché nella promozione di una politica belligerante e di conflittualità. Dicevo: l'Europa che riconosce se stessa inverando i valori della sua tradizione, che sono i valori della solidarietà e della responsabilità: i valori della solidarietà e della responsabilità: valori che evocano allora la legittimità dell'assunzione di poteri sanzionatori rispetto a chi viene meno a questi riferimenti. Penso, ad esempio, alle questioni cruciali che investono la materia dei rifugiati o dei richiedenti asilo. Abbiamo avuto, nel corso del 2016, 180.000 ingressi: evidentemente non tutti rifugiati o richiedenti asilo, ma c'era un accordo sulla ricollocazione di 160.000 cittadini. di 160.000 cittadini. Ne sono stati ricollocati circa 20.000. Ebbene, noi oggi possiamo farci forti del parere dell'avvocatura della Commissione europea,

è stata pensata ed elaborata: mi riferisco al *migration compact*, una prospettiva di cooperazione, una prospettiva che ci pone di fronte ai continenti della fame, della miseria e della sofferenza non con l'atteggiamento supponente dei nuovi colonialisti, ma nel segno della promozione di missioni civili europee.

di fronte a un fenomeno che crea problemi drammatici alle legittime aspirazioni di sicurezza dei cittadini europei, quale interpretazione diamo? Siamo in presenza di una radicalizzazione dell'islamismo o siamo in presenza di una radicalizzazione sociale e politica che viene declinata in termini islamici?

Concludo con una brevissima osservazione, che pongo come problema al collega Gozi, che so competente e sensibile. Quando si sostiene la necessità di un rapporto di cooperazione tra l'Unione europea e la NATO (nei tempi contemporanei non esiste più un pericolo di invasione dall'Est dall'Est sovietico) e quando si parla di incremento e di implementazione delle opzioni della ricerca e della capacità e si parla dell'istituzione di un fondo unico che verrebbe espunto dal calcolo delle spese ai fini del debito, si apre una prospettiva problematica. Mi domando infatti se queste risorse non possano essere calcolate e applicate ad altre materie Concludo riconfermando il sostegno alla proposta di risoluzione e, allo stesso tempo, chiedendo agli esponenti del Governo di assumere gli interrogativi che ho sollevato.

signor Presidente, signor rappresentante del Governo, noi vorremmo svolgere una riflessione di attualità. Veniamo, come tanti altri senatori, dal convegno di Farmindustria

Il Ministro però ha omesso di dire che ci è costato 3,9 miliardi e che l'unico farmaco a disposizione era un farmaco della

Dico questo perché è importante, con la legge di bilancio e di stabilità in fase di progettualità, ricordare che muoiono 15.000 persone

Tra 50 milioni e 3 miliardi e mezzo mi sembra che la differenza sia sostanziale. Questo ci fa anche riflettere sul ruolo dell'ANAC, che crediamo non serva più in Italia, perché se in se in una trattativa privata, dove si spendono 3 miliardi e mezzo (ieri abbiamo fatto una mozione sui grandi appalti della Consip e parlavamo di 2,7 miliardi), non c'è traccia di corruzione, significa che in Italia la corruzione non esiste. Con una trattativa privata, secretata e con il monopolio di una multinazionale americana,

sua richiesta, Presidente. Come già ricordato in quest'Aula, i temi che il Presidente del Consiglio si troverà ad affrontare assieme ai suoi omologhi europei rivestono un'attualità e una delicatezza particolari: le questioni investono da una parte i rapporti dell'Unione verso l'esterno (pensiamo ai temi delle migrazioni, della sicurezza e difesa); dall'altra riguardano le grandi direttrici di sviluppo interno, per sostenere e implementare posizioni comuni sull'occupazione, sulla crescita e sulla competitività. A tutto ciò si aggiunge il tema dell'avvio dei negoziati sulla Brexit: nel migliore degli scenari, sviluppi negoziali positivi consentiranno di avviare, da parte del Consiglio europeo, anche questa questione. Strettamente correlato al negoziato Brexit è il destino delle agenzie dell'Unione europea la cui sede attuale è nel Regno Unito. Unito. Sarà interessante conoscere quali modalità procedurali saranno stabilite dal prossimo Consiglio per il trasferimento di tali agenzie, anche perché il nostro Paese è uno dei futuri candidati ad ospitare la nuova sede di EMA, l'Agenzia europea per i medicinali. In particolare, saranno approvate le linee guida su cui saranno valutati i *dossier* di candidatura delle città

valuterà l'attuazione delle misure adottate per arginare i flussi migratori lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Il nostro Governo dovrà mostrarsi solido nel rivendicare gli impegni mantenuti sul fronte dell'accoglienza, dalla costruzione degli *hot spot* alla velocizzazione delle procedure di riconoscimento dei migranti; ma dovrà mostrarsi anche risoluto, a proposito della cosiddetta doppia rigidità di cui parlava il Presidente del Consiglio, nel pretendere che gli Stati dell'Unione europea rispettino gli impegni che essi stessi hanno sottoscritto, specificamente in relazione alla redistribuzione per quote dei migranti arrivati alle frontiere meridionali dell'Unione. Altra tematica estremamente attuale è quella relativa ai progressi nel campo della sicurezza esterna e della difesa. Un contesto geopolitico complesso come quello attuale, in cui le forze di frammentazione centrifuga sembrano essere prevalenti nello scenario internazionale rispetto a quelle di collaborazione solidale, richiede E chiaro che le problematiche derivanti da un quadro internazionale così convulso si riverberano anche al livello di sicurezza interna, come siamo tragicamente chiamati a testimoniare ormai quasi quotidianamente. E quindi, opportunamente, il prossimo Consiglio europeo sarà la sede appropriata per un confronto sulle situazioni interne agli Stati UE al più alto livello dei capi di Stato e di Governo. come ultimo punto delle mie considerazioni, vorrei fare riferimento ai temi dell'occupazione e della crescita. Il Consiglio europeo si è riproposto di esaminare gli sforzi finalizzati ad approfondire il mercato unico, specialmente nei settori in cui l'integrazione europea è più arretrata. Negli ultimi mesi si è rilevato da più parti, con moderata soddisfazione, che l'Unione nel suo complesso ha intrapreso una nuova strada di crescita e rilancio del lavoro. Anche l'Italia è riuscita ad invertire la tendenza di un pluriennale ciclo negativo: non abbiamo fatto sicuramente abbastanza, ed è questo il momento propizio per accelerare su questo percorso, nell'ambito di regole europee che devono essere implementate nell'ortica di sostenere gli sforzi degli Stati membri. Quindi, i *leader* approveranno le raccomandazioni specifiche per Paese e concluderanno il semestre europeo 2017. ho cercato di riassumere, è evidente che l'UE e, al suo interno, l'Italia sono chiamate, ciascuna al proprio livello, a svolgere un ruolo fondamentale di stimolo e di nuova propulsione del motore della crescita economica, della gestione del fenomeno migratorio e della prevenzione Siamo fiduciosi che il primo ministro Gentiloni Silveri sappia e possa, con il mandato di quest'Assemblea, interpretare tali esigenze presso i *partner* europei nel modo migliore e più convincente possibile.

la questione che riguarda non genericamente il rilancio dell'Europa, e anche una vera discussione sulla discontinuità con le politiche fin qui seguite dall'Unione europea. In particolare, siamo ancora dentro alla vicenda che ha fatto sì che dalla crisi

il momento di aumentare le spese per gli armamenti; dovrebbe essere invece il momento in cui soprattutto l'Italia porta avanti, all'interno dell'Unione europea, una politica contro questo tipo

Signor Presidente, il Gruppo Per le Autonomie - PSI - MAIE ha apprezzato molto l'equilibrio delle comunicazioni rese dal presidente del Consiglio Gentiloni che richiamano la credibilità delle posizioni sostenute dall'Italia sui temi oggi prioritari come la sicurezza, la lotta al terrorismo, le politiche attive nei confronti dei migranti e il negoziato sulla Brexit. Condividiamo, quindi, pienamente la linea del Governo in relazione a tali problemi. L'Italia fa infatti bene a ribadire il carattere strategico dell'Unione e a chiedere, nel contempo,

dei lavoratori, pretenda poi di continuare a beneficiare della libera circolazione delle merci. In merito alle politiche di governo del fenomeno migratorio, l'Europa deve essere più solidale, non solo a parole, ma anche con i fatti concreti. L'Italia è la frontiera d'Europa, ma finora ha operato in assenza dell'Europa, e così non possiamo certamente andare avanti. In ordine alle politiche di contrasto al terrorismo in materia di sicurezza, i Paesi europei appaiono in difficoltà dinanzi alla drammatica evoluzione che gli attentati hanno impresso.

Relativamente alla nostra espressione di voto, vorrei innanzitutto far osservare perché non accettiamo le riformulazioni proposte, essendo importante capire quali sono i punti che proprio non vanno giù ai colleghi della maggioranza.

la sinistra o il centro-sinistra! Un'altra cosa che proprio vi è indigesta è il concetto di "azioni di sostegno al reddito". Dopo aver sentito parlare di "reddito di inclusione", non mi sarei aspettato Probabilmente ciò accade perché si parla di "reddito di cittadinanza". Se volete, possiamo chiamarlo in un altro modo, ma la sostanza è che questo a voi resta molto indigesto, perché diventa impossibile mettere in atto pratiche di deflazione salariale, che è un concetto in letteratura scientifica che si pone si vuole aumentare la competitività. In realtà, non è chiaro perché in un'unione si debba competere: in unione si coopera, non si compete con la Germania, altrimenti che unione ho fatto? Faccio una divisione, al massimo. Quindi, non si capisce bene, in questo contesto, come si potrebbe essere più competitivi o più produttivi - fatto salvo che la nostra produttività è simile a quella della Germania - se non intervenendo sul salario e facendo deflazione salariale, come hanno detto autorevoli economisti. Se non puoi fare questo, devi fare deflazione.

fermo restando che uno Stato esce dagli accordi e vi entra secondo un principio di *fair play* internazionalmente riconosciuto nel corso dei secoli, per cui tanto facilmente puoi entrare e tanto facilmente poi uscire (altro concetto che evidentemente non piace). Ebbene, sul concetto del contrasto al cambiamento climatico, di cui voi non volete sentire parlare,

rischia di sparire: 50 chilometri quadrati di lago rischiano di sparire e voi riuscite a far sparire questo dall'agenda che si vuole portare in Consiglio d'Europa. Perché? Ovviamente i nostri impegni di contenimento della temperatura di 1,5 gradi possono essere fatti dalle Nazioni europee, Polonia esclusa, senza fare nulla: noi, lasciando fare, siamo in linea per ottenere

Presidente, noi ringraziamo il Governo per il parere favorevole espresso sulle nostre proposte,

necessari a chiedere il cambiamento dell'ordinamento internazionale sul salvataggio in mare, le norme del Trattato di Dublino per quanto riguarda il trattamento e il luogo dove devono stare

In realtà, di quei 39.600 ricollocamenti solo 6.500 hanno avuto luogo. Non credo che manchino all'appello soltanto la Polonia e l'Ungheria. Pertanto, il problema vero è fare davvero una politica di

essere credibili o accettabili quando in sede internazionale si chiede una politica europea comune. Noi sosteniamo

Forza Italia è tra i protagonisti, sta lavorando concretamente per dare soluzione a questi problemi. Siamo favorevoli anche alla politica europea di difesa comune.

In sintesi, ribadiamo la nostra richiesta al Governo di difendere con determinazione gli interessi italiani in sede internazionale e, in particolare, di tenere fede agli impegni che assume accettando le nostre richieste, in particolare sulla politica migratoria, sulla sicurezza, sulle questioni economiche e sulle sanzioni alla Federazione russa che parecchio danneggiano la nostra economia.

sono d'accordo con il giudizio di fondo che ha dato il Presidente del Consiglio sulla situazione dell'Unione europea, e cioè sul fatto che si è ripartiti e non ci si arresi o rassegnati, né c'è stato un crollo. Bisogna cambiare e andare avanti.

europea e altre come la nostra che ritengono che il destino presente e futuro sia di stare nell'Unione europea, ma che l'Unione europea debba e possa essere cambiata. Questo è un punto per noi fondamentale.

riforma e il cambiamento dell'Unione europea. A me pare questo un punto decisivo e in fondo quello che caratterizza l'attuale maggioranza di Governo.

ringrazio Alternativa Popolare per il fatto di non avere ambiguità rispetto a questo punto. È fondamentale ancorarsi alla prospettiva della costruzione dell'Unione europea.

E capisco le difficoltà del senatore Candiani, che registra le sconfitte del lepenismo, di parlare d'altro. Noi abbiamo posto le questioni di una stretta connessione tra riforme democratiche e riforme economico-sociali.

le politiche che ci spettano nei confronti dei nostri vicini e dare sicurezza ai nostri cittadini all'interno dell'Unione. L'ultima parola riguarda la situazione dei migranti.

se vogliamo solidarietà dall'Europa - e la vogliamo - dobbiamo pretenderla anche dall'Italia, perché tutti i Comuni che non accettano chi ha diritto all'asilo (e si

**Il Senato non approva.**